coloro che sono intervenuti. Devo però dire che è stato un dibattito poco incentrato sulla manovra e molto sugli emendamenti. Credo che questo debba essere rivisto. Voglio quindi partire dal dibattito sulla manovra per poi passare agli emendamenti. Il dibattito sulla manovra non può che essere positivo, perché non possiamo non rivendicare il suo carattere espansivo. Una manovra Una manovra che punta al rilancio di questo Paese e che cerca di rendere più forti i segnali di ripresa che ci sono.

Un Paese che vedeva un prodotto interno lordo con il segno negativo e, ora, un prodotto interno lordo con il segno positivo. Un Paese che continuava a perdere posti di lavoro e che si ritrova adesso

valutare la manovra nel suo complesso e apportare quelle che possono essere modifiche utili per il Paese. E di queste ne troviamo davvero tante.

nell'applicazione della legge di bilancio, forse un compito per la prossima legislatura sarà proprio quello di ridefinire le regole su come affrontare la legge di bilancio. Penso che quello del Parlamento sia un ruolo complessivo, di Camera e Senato. Il Senato ha fatto una parte,

abbiamo fatto quel che dovevamo per il Paese ovvero abbiamo concentrato nel poco tempo a disposizione tutto il lavoro che dovevamo fare

altro aspetto importante che vorrei sottolineare è il grande lavoro che è stato fatto da molti senatori

voglio ringraziare qui chi ha lavorato in modo disinteressato e con grande generosità per arrivare a questi testi condivisi. In particolare, ne cito uno solo per ringraziare tutti. È il senatore Angioni, che ha lavorato moltissimo per arrivare a soluzioni condivise: e qui lo ringrazio. Abbiamo fatto provvedimenti importanti che qualche volta le opposizioni hanno citato, secondo me, nella *verve* di una campagna elettorale che ormai è partita, ma sui quali proverei a fare una piccola riflessione. In modo un po' svilente qualcuno ieri, non ricordo neanche chi, ha detto che abbiamo dato contributi a manifestazioni carnevalesche, con una leggera sfumatura dispregiativa. Io vorrei ricordare che i carnevali di Venezia, di Viareggio, di Sanremo, di Ivrea e tanti altri che non ricordo e non voglio citare, sono grandi manifestazioni che portano al territorio lavoro, turismo e danno impegno per tutto un anno di lavoro. Io cito il mio territorio: Io cito il mio territorio: a Pinerolo, quando c'è il carnevale, arriva un sacco di gente e lavorano tutti. Io credo che, all'interno delle manifestazioni culturali, tutte queste cose debbano avere la loro dignità, anche quando sono più orientate al settore del turismo e ad alimentare, comunque, la nostra economia.

il grande intervento fatto sull'università e sui ricercatori, sul quale tutti erano concordi nel dire che dovevamo lavorare, perché per noi questo è un settore strategico, perché i nostri giovani devono rimanere a pensare qui e devono lavorare qui. Quindi - ripeto - questo è un settore strategico. Abbiamo citato le pensioni, un intervento importante a favore di lavoratori che rappresentano le categorie più indifese, che hanno fatto per tutti noi i lavori più faticosi e ai quali dobbiamo riconoscere questo impegno. Ricordo l'assunzione, soprattutto, di un principio, di un riconoscimento sui *caregiver*, cioè sulle persone che nelle famiglie assumono l'impegno di occuparsi dei propri familiari, anche a discapito della propria vita, del proprio lavoro e delle proprie potenzialità di vita.

per effetto del femminicidio e che si ritrovano davvero da soli: da un lato, perdono la madre e, dall'altro, si ritrovano senza il padre. il padre. Questo è stato un passaggio importante della Commissione, perché tutta la Commissione, unanimemente, ha riconosciuto che l'impegno in questa direzione era un impegno da assumersi ora e non più procrastinabile.

ricordo lo stanziamento in favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, che è un intervento piccolo, ma comunque significativo di un'attenzione a nostri concittadini con difficoltà.

Ringrazio il Presidente della Commissione, perché davvero, anche lui, con tanta pazienza, ha cercato di rispondere alle esigenze di tutti, anche quando queste erano contrapposte, cercando una giusta mediazione. Ovviamente ringrazio il mio correlatore, perché abbiamo combattuto insieme questa battaglia. Ringrazio i senatori presenti, che hanno, comunque tutti, anche le opposizioni, condiviso con noi questo percorso e hanno

il lavoro complessivo della Commissione, non fermarci a metà, per cui solo quelli che erano stati fortunati e che erano capitati nella prima parte del dibattito trovavano ristoro. Ci sono

Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, gli uffici di tutti i settori che si sono impegnati con noi, in modo particolare ovviamente quelli del

la mia collega è già stata abbastanza esaustiva e la ringrazio anche per l'amicizia e la pazienza che hanno avuto nei miei confronti, per il grande lavoro e per il contributo che ha dato. Vorrei essere molto rapido nel dire che ho avuto la fortuna di avere in Commissione colleghi sensibili ai temi posti dal Governo. Ho riscontrato grande attenzione.

Devo ringraziare personalmente anche il vice ministro Morando, che con poche risorse ha fatto le magie per venire incontro alle richieste dei gruppi.

società con scopo di lucro, potendo avere un futuro nel campo sportivo anche a livello privatistico. Ringrazio fortemente i miei colleghi, il Governo e la mia collega relatrice

credo che sia necessario, ora che stiamo per decidere, tornare sulla struttura di fondo di questo disegno di legge di bilancio su cui il Senato sta per pronunciarsi. I pilastri fondamentali di questo provvedimento sono tre: il primo è rappresentato dalla scelta di ridurre di 15 miliardi di euro la pressione fiscale, prevista a legislazione vigente, nella convinzione che un così forte aumento dell'imposizione indiretta, IVA e marginalmente accise, avrebbe messo a rischio la ripresa economica che si viene finalmente consolidando. Il secondo pilastro è confermare e rafforzare ulteriormente il forte sostegno in atto già nel 2017 agli investimenti privati, nella convinzione che si possa, per questa via, favorire quel recupero di produttività del lavoro e dei fattori che è indispensabile per recuperare capacità competitiva nel contesto dell'economia globale.

perché senza questo rafforzamento rischia di rimanere indietro rispetto al fattore capitale nel tumultuoso procedere di globalizzazione per un verso e rivoluzione tecnologica per l'altro che si stanno sostenendo reciprocamente nel determinare cambiamenti sconvolgenti nell'assetto dell'economia globale. questi tre pilastri fondamentali tale struttura fondamentale viene pienamente confermata ed è facile arrivare a questo giudizio obiettivo e difficilmente contestabile,

uno. Bisogna dedurre quindi che l'intero Senato, maggioranza e opposizione, ha deciso che questi tre pilastri fondamentali rimanessero intatti,

Dopo avere detto ciò, c'è un'ulteriore constatazione da fare: nessun emendamento - ripeto nessun emendamento su 4.000 è orientato a ridurre la portata dei tre pilastri, cioè a utilizzare parte delle risorse dedicate

la capacità finanziaria, utilizzando cioè una quota delle risorse relative alla riduzione della pressione IVA, prevista a legislazione vigente, interventi sul fattore del sostegno all'investimento privato e a interventi a sostegno del fattore lavoro, specie nella sua componente giovanile. Nessun emendamento di utilizzare almeno una quota delle risorse dedicate a tale scopo per finanziare altri tipi di attività e proposte. Quindi, dobbiamo dedurre che, consapevoli di questa intangibilità della struttura essenziale della legge di bilancio, maggioranza - e questo è abbastanza ovvio - ma anche anche opposizione - ciò è decisamente meno ovvio - hanno concentrato la loro attenzione, cioè le loro proposte emendative, sulle componenti non essenziali dell'edificio costituito dalla legge di bilancio al nostro esame. Questo non è il giudizio di parte del Governo; è un giudizio che trova alimento nell'esame puntuale degli emendamenti presentati alla nostra discussione. Le opposizioni hanno, dunque, rinunciato - il mio giudizio è che abbiano fatto bene, ma questa non è più una valutazione oggettiva - a presentare per il dibattito addirittura

di fondo che, invece, avevano caratterizzato le risoluzioni parlamentari sulla Nota di aggiornamento al DEF, che sia Forza Italia e Lega, da una parte, sia Movimento 5 Stelle, dall'altra, hanno presentato alla nostra discussione proprio soltanto qualche settimana fa.

in quanto rappresentante del Governo che deve misurarsi con le proposte emendative, sulla riforma strutturale introdotta in via di fatto per il dibattito parlamentare del Senato sulla legge di bilancio con l'utilizzazione della fase di illustrazione per ottenere al Senato lo stesso risultato concreto che si ottiene alla Camera in forza di Regolamento attraverso la procedura della segnalazione ufficiale da parte dei Gruppi degli emendamenti che essi intendono sottoporre davvero alla discussione. Si tratta

un emendamento in materia di pensioni di Forza Italia e Lega che traducesse in proposta legislativa l'indicazione assolutamente fondamentale nella risoluzione sulla Nota d'aggiornamento al DEF di Forza Italia e Lega volta a riportare la regolazione in materia di pensioni in Italia alla situazione pre-Fornero. Sia i senatori della Lega che quelli di Forza Italia sanno che non sto parlando di una cosa che mi sto inventando in questo momento. Nella risoluzione di Lega e Forza Italia era presente questa indicazione e, dato l'enorme rilievo finanziario che questa indicazione ha, io mi aspettavo che con la necessaria copertura questa indicazione si traducesse in un emendamento parlamentare. Bene, questo emendamento non c'era al nostro esame, che le stesse forze proponenti assegnano a questa proposta per il futuro del Paese: la fanno, l'hanno fatta durante la risoluzione della NADEF, ma è patente che non ci credono; se ci avessero creduto, l'avrebbero presentata come proposta emendativa alternativa alle soluzioni indicate nella legge di bilancio. Così come, per la prima volta, ho cercato invano tra gli emendamenti segnalati l'emendamento del Movimento 5 Stelle volto ad introdurre in Italia il reddito di cittadinanza, una misura che vale appena un po' di più in termini finanziari di quella che viene introdotta nella legge di bilancio volta a eliminare l'aumento di pressione fiscale IVA che è disposto dalla legislazione vigente a partire dal 1° gennaio del 2017. Per valutazioni tecniche condivise tra il Governo e il Gruppo del Movimento 5 Stelle, l'introduzione di un reddito di cittadinanza, così come disegnato dal Movimento 5 Stelle, vale grosso modo 17 miliardi di euro; allo stesso

di bilancio - delle cosiddette clausole di salvaguardia, cioè degli aumenti di IVA previsti a legislazione vigente, vale circa 15 miliardi di euro. Quindi sarebbe stato legittimo proporre l'una cosa al posto dell'altra; grosso modo sarebbe stata una soluzione alternativa. Non è stata presentata questa proposta, né ne sono state presentate altre, il che vuol dire che evidentemente si sta ragionando sopra l'esigenza di "trovare" rispetto al passato coperture finanziarie più solide rispetto a quelle che tradizionalmente vengono poste a copertura di questo provvedimento. Mi sembra quindi di avere segnalato un fatto, quello che riguarda l'assenza della proposta fondamentale e alternativa sia del Movimento 5 Stelle sia di Forza Italia e Lega Nord, che può essere giudicato positivamente o negativamente, ma è difficile negare che sia un fatto. è a partire da qui naturalmente che a me sembra che si debba ragionare delle implicazioni politiche generali della proposta di legge di bilancio al nostro esame. Fin qui le considerazioni di ordine generale. Venendo invece alle misure concretamente introdotte, ferma la struttura fondamentale della legge di bilancio considerata intangibile sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, le modifiche introdotte introdotte ai margini, anche se si tratta di modifiche consistenti, durante la lettura della Commissione bilancio del Senato della legge, sono in questo contesto assolutamente significative. La prima innovazione è rappresentata dalla traduzione in legge

Sono molto contento dell'attenzione che riesco a ottenere, soprattutto dal Gruppo del Partito Democratico, ma lasciamo perdere. della traduzione in legge del contenuto dell'accordo concluso tra il Governo e due delle tre organizzazioni sindacali in fatto di regolazione del sistema previdenziale pubblico. Insisto sul valore politico di questo fatto non solo e non tanto in sé, perché si tratta di un intervento che sotto il profilo del rilievo finanziario è significativo, ma non incidente come lo sono state le misure in materia di pensioni che abbiamo via via adottato a partire dal 1995 in poi, sotto la direzione e l'impulso di Governi diversi che tuttavia, per l'essenziale, hanno sempre agito in coerenza con l'obiettivo di stabilizzare la spesa previdenziale e di ridurre le enormi sperequazioni che caratterizzavano il sistema previdenziale pubblico prima di quella data. Mi riferisco esplicitamente - per essere chiaro - all'intervento del Governo Dini del 1995, all'intervento successivo del Governo Prodi

È chiaro che l'intervento di cui stiamo parlando ora in materia di pensioni non ha nemmeno lontanamente l'incidenza, sia finanziaria che effettiva, sulla regolazione del sistema di questi interventi che ho richiamato. Tuttavia, l'intervento segna una sistemazione ai margini molto rilevante, perché finalmente codifica e crea le condizioni per una codificazione assai più significativa e definitiva (per quanto possa essere definitiva la scelta in questo campo) dei cosiddetti lavori usuranti, e per ora gravosi. sono naturalmente, per loro definizione, particolarmente complessi in un'economia che continua a cambiare e quindi produce sistematicamente, da un lato, per fortuna, grazie alle nuove tecnologie, la fuoriuscita di categorie di lavoratori da quelle attività lavorative e che presentano la caratteristica di accorciare l'attesa di vita al momento del pensionamento ma, dall'altro lato, la stessa rivoluzione tecnologica introduce nuovi rischi sotto questo profilo per altre altre categorie di lavoratori. Se quindi l'economia ha questa caratteristica, non smetteremo mai di aggiornare questo elenco sia per escludere sia per includere categorie di lavoratori, ma non c'è dubbio che qui c'è qualcosa di nuovo, strutturale e significativo che viene introdotto da questa modifica alla regolazione del sistema previdenziale rispetto alla fase precedente. Ciò che però rileva sul piano politico è il recupero pieno di una relazione - non importa poi che l'esito abbia visto due organizzazioni sindacali convergere con la proposta del Governo e un'organizzazione sindacale invece giudicarne negativamente gli esiti: la dialettica continuerà a svilupparsi - tra Governo e parti sociali

secondo aggiustamento significativo ai margini è l'introduzione della *web tax*, una novità importante a mio parere mediamente sottovalutata dal dibattito. L'Italia prende l'iniziativa, rompe gli indugi, in un contesto internazionale che su questo punto sta modificando i suoi orientamenti.

dovuto pensare, per interessi nazionali contrapposti, di menare il cane per l'aia per molto tempo perché, sulla base di una elaborazione ormai matura, se la soluzione di dimensione europea ed internazionale non fosse venuta immediatamente, l'Italia avrebbe preso l'iniziativa di introdurre la cosiddetta Non è arrivata la soluzione; è venuta la soluzione elaborata, in sede parlamentare - e ciò la rende ancora più significativa e vorrei ringraziare il senatore Mucchetti a questo proposito

mi scusi, signor Presidente, prenderò qualche minuto in più, se me lo concede - della particolare e significativa richiesta di aiuto che con questa soluzione rivolgiamo al sistema bancario italiano. Voglio dirlo in questa replica con chiarezza. Sappiamo che senza il contributo del sistema bancario e degli intermediari finanziari la *web tax* che abbiamo delineato non avrebbe potuto funzionare (per questo non abbiamo esitato a introdurre l'ipotesi del sostituto di imposta per la concreta esazione di questa tassa altrimenti non esigibile), ma siamo pronti ad un confronto con gli istituti bancari per trovare le forme di una compensazione, perché sappiamo che gli abbiamo dato da svolgere un ulteriore Lo faremo certamente sviluppando un confronto aperto e trasparente, alla luce del sole, con le rappresentanze di questi istituti.

con un'aggiunta molto significativa di risorse rivenienti dall'articolo 92, il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, per un intervento a favore della famiglia, in particolare della natalità. Si tratta di un intervento già finanziariamente molto significativo e che se dovrà essere aggiustato alla Camera lo sarà, perché il Governo condivide la scelta, in particolare avanzata dal Gruppo AP, di sostenere questa prospettiva con concrete e puntuali riforme da introdurre nel corso dell'esame di questo disegno di legge di bilancio. Un altro intervento intervento da realizzare in cooperazione con le Regioni è rappresentato dalla proposta di introduzione di una norma che riguarda la cooperazione tra Regioni e Stato centrale per la riduzione riduzione dell'impatto sociale del cosiddetto *superticket* in sanità. Un volume significativo di risorse è stato dedicato all'introduzione di una di una cooperazione, appunto, tra Regioni e Stato centrale su questo versante. Un ultimo, a mio avviso, significativo intervento riguarda invece la spesa in conto capitale, e cioè l'intervento sul cosiddetto quadrilatero Umbria-Marche, volto finalmente a

La lettura della Camera potrà completare questo disegno attraverso l'introduzione, in particolare, di misure sul versante delle autonomie regionali e locali: le Regioni a statuto ordinario e il completamento delle operazioni realizzate sul versante delle Regioni a statuto speciale. Penso in particolare

alla Camera perché là ci saranno le risorse recate dal decreto fiscale (attraverso l'approvazione di uno specifico emendamento che il senatore Laniece ben conosce). Infine, alla Camera bisognerà accompagnare la rivoluzione - perché di questo si tratta - dell'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria anche per le transazioni commerciali tra privati, con misure specifiche e contemporanee di riduzione degli adempimenti, quindi quindi con un aumento delle semplificazioni degli adempimenti fiscali in carico ai contribuenti. Se vogliamo consolidare la novità difficilmente sopravvalutabile dell'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria anche per le transazioni commerciali tra privati, se vogliamo dimostrare che funziona, bisogna che i contribuenti non ricevano semplici promesse che sarà semplificato il sistema, ma vedano la semplificazione del sistema procedere contemporaneamente all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria. A queste condizioni, sarà un successo e sarà un'innovazione decisiva nella battaglia per la riduzione della pressione fiscale in Italia. Presidente, vorrei sottoporle due questioni di natura regolamentare.

contezza nelle ore recenti, e a votare gli emendamenti. Diversamente, non so come potremo rispettare il Regolamento del Senato. Capisco che la fiducia sia stata annunciata in maniera irrituale, già in Commissione bilancio, ma non possiamo dare per scontato che i lavori dell'Assemblea si debbano interrompere in attesa di un qualcosa che formalmente non è stato annunciato. Le chiedo conferma di questo, dopodiché eventualmente,

Signor Presidente, come ricordava il collega Endrizzi, il Governo ha preannunciato in sede di Commissione bilancio l'intenzione di porre la questione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione. Com'è noto, moltissimi sono stati gli emendamenti accolti, anche praticamente nella mattinata di ieri, il che richiede un supplemento di lavoro da parte della Ragioneria generale dello Stato nella definizione e nel controllo dell'elaborato. Trattandosi di un lavoro particolarmente complesso e laborioso,

nuova finestra"). Salutiamo gli alunni, le alunne, gli accompagnatori e i docenti dell'Istituto comprensivo «Via Val Maggia» di Roma, che seguono i nostri lavori.

riconosce, richiama e fa propria. Voglio dire che la legge di contabilità prevede che non siano ammissibili emendamenti che non abbiano impatto sulla finanza pubblica. Non sono ammissibili emendamenti, parti di emendamenti o vere e proprie leggi con contenuto ordinamentale La legge di bilancio non è la discarica delle responsabilità del Governo, di tutte le cose che il Governo non è riuscito, non ha voluto o non ha potuto realizzare e di quelle che ha dovuto pagare ai soci della prossima campagna elettorale in termini di marchette localistiche; anche queste sono chiaramente escluse dalla legge di bilancio. *(Applausi dei senatori

dalle sue responsabilità in termini di principio e poi le motiverò perché faccio richiamo ad esse. Il Regolamento del Senato, al Capo XV, dedica uno spazio rilevante e dettagliato alla procedura di esame degli atti attinenti al bilancio dello Stato, affidando al Presidente del Senato, cioè a lei, Presidente, quale garante del rispetto della legislazione vigente in materia di contabilità e del Regolamento stesso, il compito, ad esempio, già prima dell'assegnazione, di accertare l'eventuale presenza di disposizioni estranee. E lei lo ha esercitato, questo compito, se ne è assunto la responsabilità

a queste normative, in questa sede, un rango sovraordinato alla legge di bilancio stessa. Non può la legge di bilancio violare il Regolamento e ciò che il Regolamento tutela.

Come ho detto prima sia le questioni localistiche, sia quelle prive di rilevanza ai fini del bilancio sia quelle meramente ordinamentali sono escluse; tale esclusione è prevista dal Regolamento, e di questo Regolamento lei è il principale garante, insieme alla Giunta per il Regolamento. le norme introdotte in maniera furtiva e in violazione del Regolamento? Ne citavo solo alcune, ma è veramente un *pot-pourri:* il contributo in favore dell'Accademia Vivarium Novum, i contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo, il fondo per la conservazione e l'informazione degli archivi dei movimenti politici,

Poi abbiamo gli interventi per il Comune di Cogoleto e via dicendo. Sono stati anche richiamati molto dettagliatamente dalla collega Montevecchi non più tardi di ieri sera. Se guardiamo poi agli emendamenti di iniziativa del Governo, troviamo il grande progetto Pompei, il personale ATA delle scuole, il settore aerospaziale, le modifiche al piano scuole belle. Non permetto speculazioni su questo punto. Non siamo a discutere del merito e della bontà di queste norme ma, come è già stato detto, del fatto che esse vengano sottratte ad un dibattito parlamentare e essere discusse in queste sedi seguendo la procedura corretta, cioè nel rispetto del Regolamento. Abbiamo poi altri emendamenti d'iniziativa parlamentare, come le modalità d'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, del senatore Santini, o l'attribuzione di funzioni sui rifiuti all'Autorità

la legge di bilancio fu assegnata al Senato, che queste materie non rientrino nel rispetto della legge di contabilità.

fin d'ora, sulla base del testo A, a maggior ragione se verrà posta la questione di fiducia sul maxiemendamento, la invito ad assumersi una responsabilità che è solo sua.

tutta la responsabilità passa al Presidente della Commissione che ha lavorato. Ritornerò nelle mie prerogative non appena ci saranno gli emendamenti e si tornerà in Aula. Questo è il Regolamento;

Signor Presidente, aspetto un attimo perché il senatore Sposetti ha preso l'abitudine di interrompermi sempre sia in Commissione, che in Aula. Molto divertente. Finito? Bene. Volevo solo fare una notazione di fronte a questo spiacevole episodio. Tante volte è successo che il maxiemendamento non fosse pronto e quindi la cosa non mi sconvolge più di tanto; magari si poteva prendere qualche precauzione nella maggioranza o si facevano più interventi, almeno per salvare la forma.

alle quali non abbiamo risposto mai - parlo delle opposizioni nel loro complesso - con atteggiamenti, non dico ostruzionistici, ma anche di semplice rispetto di banali regole di procedimento, come ad esempio votare tutti gli emendamenti o cose del genere. C'è stato un dibattito, dibattito, una chiusura totale nei confronti degli emendamenti delle opposizioni, ma di questo parleremo. Vorrei altresì rilevare che ho sentito sia da parte della relatrice che da parte del Governo sottolineare, quasi come se fosse elementare, il fatto che la legge sia fatta a rate, una al Senato e una alla Camera, così come avvenuto peraltro per il

sia uno schiaffo anche a noi nel nostro ruolo di rappresentanza perché noi, a Costituzione vigente, siamo tenuti, oltre ad averne il desiderio, ad esaminare tutte le leggi che passano con una lettura piena e non solo con un voto di fiducia su un testo acquisito da un'altra Camera.

detto di non aver notato che erano stati presentati emendamenti che configuravano un'impostazione di manovra diversa, finalmente prenderebbero coscienza

prodotta nei Gruppi una situazione difficile a causa del preannuncio stesso del voto di fiducia, che poi come vediamo oggi non si è in grado di formalizzare rapidamente, visto che il maxiemendamento non è ancora pronto. Credo però

oggi c'è un problema degli Uffici nel poter fascicolare gli emendamenti che sono stati presentati e quindi, anche volendo, in questo momento non siamo in condizione di andare avanti nella procedura è il problema che abbiamo, proprio per le questioni che lei ha rappresentato.

preso Signor Presidente, lei ha rappresentato un quadro abbastanza chiaro: la sua responsabilità si manifesta, si realizza, si concretizza nel momento in cui il testo arriva in Aula.

già disponibile, o prossimo ad arrivare, ed è su quel testo che io richiamo la sua responsabilità.

a valutare sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale e di contenuto, nonché sulla presenza al suo interno dei milleproroghe, che già di per sé sono una vergogna istituzionale e costituzionale in quanto ledono l'affidamento

nel merito non voglio nemmeno discutere, ma, con riferimento alla correttezza regolamentare, lei, su questo testo A, è chiamato a rispondere. E sarà chiamato nuovamente nel momento in cui il Governo presenterà il maxiemendamento. Se avverrà, perché io sui fantasmi non sono abituato a ragionare.

Presidente, intervengo per annunciare ai colleghi che il maxiemendamento bollinato è in fase di trasmissione e, proprio per riguardo nei confronti dei colleghi e ricordando anche il ritardo di una delle ultime fiducie,

pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo degli articoli della Parte I - Sezione del disegno di legge n. 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che recepisce le modifiche approvate dalla Commissione con alcune correzioni e integrazioni di carattere tecnico e istituzionale.

l'ammissibilità delle parti del testo A, e ora del maxiemendamento, rispetto ai vincoli imposti dalla legge di contabilità per quanto riguarda la legge di bilancio; vincoli che - lo ricordo - sono confermati

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo della Parte I - Sezione I del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2018. Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti trentacinque minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. La chiama avrà pertanto inizio intorno alle ore 18. Dopo il voto di fiducia si passerà alla votazione degli emendamenti e degli articoli della Parte II - Sezione II del disegno di legge. La seduta sarà successivamente sospesa per consentire al Governo di presentare la Nota di variazioni al bilancio che, non appena trasmessa, sarà immediatamente deferita alla 5ª Commissione permanente. L'Assemblea procederà quindi al voto della Nota di variazioni e alla votazione finale del disegno di legge di bilancio con procedimento elettronico. Le dichiarazioni di voto finali si svolgeranno in un'unica fase, coincidente con le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia. È stato stabilito per le ore 19 di venerdì 1° dicembre il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di riforma organica del Regolamento del Senato,

*(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla fine è arrivato anche il maxiemendamento. Un parto difficile, ma alla fine avete generato il vostro mostriciattolo. Malgrado l'attesa, e malgrado l'ennesima fiducia, oggi sarà una bella giornata, una splendida giornata, come diceva il grande Vasco, perché finalmente sarà l'ultima, o la penultima di una serie infinita di fiducie. Siete al capolinea, cara Ministra. *Fini la musique*. Mi voglio rivolgere ai colleghi del Partito Democratico e a coloro che in quest'Aula hanno sulla coscienza un numero abnorme di fiducie:

A tale proposito, colleghi, io vi inviterei a rileggere cosa dichiarò il 24 febbraio 2014, proprio in quest'Aula, il neo presidente del Consiglio Renzi Matteo. Nel chiedere la prima fiducia di una lunghissima serie, che oggi dovrebbe chiudersi, apostrofava l'Assemblea del Senato con la sua inconfondibile arroganza, ricordandoci che la fiducia è una cosa seria, che dare la fiducia al suo Governo era una sorta di privilegio per questo Senato, sentenziando, e cito: «oggi la fiducia significa proporre una visione audace, unitaria e per qualche aspetto innovativa, che parte dal linguaggio della franchezza con il quale comunico fin dall'inizio» lui comunicava, Renzi ci comunicava

Tutti noi ricordiamo quei momenti nei quali, con prodigiosa disinvoltura, Matteuccio vostro ha raggirato e ingannato gli italiani. Sicuramente un parolaio da Nobel.

la prima volta che l'avete chiesta agli italiani, vi hanno rispedito al mittente. Vi ricordate il *referendum* sulla riforma costituzionale? Ma veniamo al provvedimento sul quale chiedete la novantesima fiducia: la legge di bilancio. Non ci aspettavamo i miracoli, ma almeno il minimo sindacale. Una legge di bilancio dovrebbe dare impulso all'economia, rinvigorire il sistema produttivo, stimolare l'impresa, dare un'iniezione di fiducia al mercato. Ridare fiducia e speranza agli italiani: questa è l'azione che tutti i Governi cercano di sostenere a favore del proprio sistema economico e sociale. Nulla di tutto questo. Tutto in linea con il disastro generato in questi anni.

del Gruppo della Lega hanno visitato le zone terremotate. Bene, anzi male. Quello che tragicamente si vede è il risultato del vostro Governo: un abbandono sconcertante, macerie e desolazione. è la rappresentazione plastica del vostro Governo, che è uguale alle zone terremotate che avete abbandonato. A tal proposito, è sempre e comunque opportuno ricordare di nuovo le parole di quel famoso 24 febbraio e sempre di quel famoso Renzi Matteo, in questo in questo caso accompagnato dall'illustre collega nonché archistar Renzo Piano, che definirei in questo caso candido ispiratore, correo però di voler pretendere da Matteo Renzi l'impossibile. Ovvero che la sua affermazione, o invito da parte di Renzo Piano, a rammendare i nostri territori e le periferie, non producesse nella testa di Renzi un'interpretazione bovina e alla lettera del pensiero, accademicamente senza inibizioni, di Renzo Piano, male interpretato però da Renzi. Cari colleghi, Renzi ha infatti lavorato di toppe, un po' come faceva mia nonna regolarmente con i miei pantaloni quando ero ragazzino, con la differenza che le toppe di Matteo Renzi e le vostre sono peggio del buco, come questo bilancio. La vostra è un'azione rattoppata, fatta di rimedi momentanei e disarticolati. In questi anni, partendo dal Governo Monti, abbiamo assistito ad un esponenziale aumento della pressione fiscale, che avete sempre giustificato affermando che

Ma alla storia, ahimè, passerà per colui che ha fatto una legge che porta il suo nome, appunto la legge Delrio, distruggendo le Province e creando il caos politico e amministrativo in territori amministrati in maniera eccellente, con criterio e giudizio. inoltre, decisioni rimandate, come quelle sull'accordo con la Confederazione elvetica, che mi sta particolarmente a cuore e che interessa 90.000 lavoratori transfrontalieri, ed è fermo da due anni; fermo da due anni; 90.000 lavoratori nell'incertezza, con la sicurezza che quell'accordo comunque va riscritto. La lista delle vostre malefatte è infinita, ma c'è una questione che è insostenibile. Il nostro Paese continua a detenere il primato dell'*import* dei clandestini e dell'*export* dei giovani che lasciano il nostro Paese. Colleghi, sulla questione va fatta una seria riflessione. Attenzione, stiamo perdendo un'intera generazione sulla quale dovremmo invece fondare il nostro futuro. I nostri giovani lasciano un Paese nel quale non vedono prospettive, un Paese che non dà né speranze né - ripeto - prospettive. La notizia è di oggi:

Oggi i giovani che lasciano il nostro Paese non sono più quelli riconducibili alla definizione di Max Frisch «volevamo braccia, sono arrivati uomini». Stiamo perdendo una moltitudine di professionisti, di tecnici, di gente altamente qualificata. Siamo già passati da quelli del primo impiego ai professionisti di altissima qualità.

Con chi stiamo sostituendo gli italiani che lasciano il nostro Paese? Voi credete che sia giusto ciò che sta accadendo? La cosa più demenziale e insostenibile è che i nostri *partner* europei, caro Ministro, patrocinati dalla matrigna Europa, sono lesti a chiudere le frontiere a Ventimiglia o al Brennero, anche con i carri armati se dovesse servire. Invece noi favoriamo questa invasione incontrollata, per poi chiudere in bellezza

affermando che di una cosa siamo certi a proposito della presentazione del conto. Siamo al capolinea e il conto sulle vostre malefatte ve lo presenteranno gli italiani a marzo, quando finalmente anche nel nostro Paese avremo elezioni libere e democratiche; allora forse capirete. Signor Presidente, colleghi, sapevamo che sarebbe stata posta la questione di fiducia sulla legge di bilancio, non è la prima volta, credo che siamo alla quinta, ma per me non è questo il problema.

Ci sono anche risposte a degli emendamenti presentati da colleghi, che forse sono risposte un po' troppo soggettive e troppo univoche, in qualche modo, e questo non l'ho molto condiviso.

Presidente, in questa legge di bilancio il Governo esce allo scoperto in difesa delle multinazionali dell'azzardo. Non bastava il rinnovo senza gara della concessione del gratta e vinci nel decreto-legge fiscale. Ricordo che quel rinnovo senza gara contrasta con i principi delle nostre normative sui contratti pubblici, contrasta con le disposizioni europee in materia di concorrenza, perché senza gara viene rinnovata una concessione, di fatto monopolistica, quando era prevista la possibile assegnazione a quattro soggetti diversi. Rinunciando ad una gara, il Governo si rende responsabile di un possibile danno erariale. Ma c'è un valore più ampio da tutelare: la trasparenza su una materia sensibile sia sul piano sociale che finanziario. Stiamo parlando del gratta e vinci, gli innocui gratta e vinci; sono azzardo a bassa latenza, cioè ad alto potere di dare dipendenza, perché tra la puntata e l'esito passano pochi secondi e si genera così una alternanza di fasi emotive che risucchiano nella coazione a ripetere. Ma lo sapete

ai giovani? E poi ci sono gli anziani: sapete quanti si svenano con i gratta e vinci? In questa Aula qualcuno sa che sono stati messi in vendita apparecchi appositi per grattare automaticamente i tagliandi? Ognuno di voi, se nella vita reale apre gli occhi, dentro un punto vendita può vederle queste cose. E su questo disastro sociale si offre un affare miliardario per Lottomatica, una società che ha trasferito all'estero la sua sede ma è stata molto generosa con i partiti italiani. Non bastava tutto ciò; il Governo in questa legge di bilancio concede il *bis* e mette nel mirino le leggi regionali e i regolamenti comunali, come quelli di Torino e Roma, che vietano l'offerta di azzardo vicino a chiese, scuole, luoghi sensibili. Sappiamo infatti che la facile accessibilità, direttamente nei luoghi di vita e aggregazione, facilita il precoce inizio dell'azzardo: ce lo troviamo sotto il naso ovunque. E iniziare precocemente significa aumentare il rischio di dipendenza e in forme mediamente più gravi. L'esplosione dell'azzardo di massa è andata di pari passo con la liberalizzazione selvaggia; e con questa sono aumentati gli affari anche per le mafie. Queste norme contrastano questi fenomeni, si sono rivelate efficaci nel proteggere la popolazione e perciò sono invise alle concessionarie del settore, malgrado tutelino i cittadini. Mesi fa il sottosegretario Baretta contestò che se allontaniamo l'azzardo da chiese e scuole, c'è il rischio che si formino delle isole di azzardo, dei quartieri a luci rosse. Proprio così. così. È lui stesso quindi ad accostare l'azzardo alla prostituzione e al degrado. Sia dunque coerente e lo ammetta: almeno vicino a scuole, chiese e luoghi frequentati da fasce deboli l'azzardo non ci può stare. Invece no: in legge di bilancio, all'articolo 90, il Governo afferma che la necessità di svolgere le gare per le nuove concessioni sulle scommesse (dunque, c'è scritto anche qui che le gare bisogna farle),

Proroga le concessioni in essere e obbliga le Regioni ad adeguare le proprie leggi sulla dislocazione dei punti di azzardo, secondo l'intesa raggiunta il 7 settembre in Conferenza unificata. come dovrebbero adeguare le proprie leggi? Questo non è per niente chiaro. Il punto 5 dell'accordo prevede una clausola di salvaguardia in materia di prevenzione e contenimento dell'azzardo, riferita però ad alcune specifiche azioni di contrasto: le Regioni che hanno leggi più restrittive in questo campo potranno mantenerle. Anche le altre potranno adottare misure più efficaci, se necessario. Ma - appunto - la clausola si trova al punto 5; le distanze minime da scuole, chiese e luoghi sensibili sono trattate invece, separatamente, al punto 2, dove nessuna salvaguardia è prevista. Anzi, è stato inserito un Regioni ed enti locali «nel tutelare la salute» debbono tenere conto degli investimenti privati e non possono, con leggi e piani urbanistici, determinare zone libere dall'azzardo. Inspiegabile è la leggerezza nell'accettare questo pasticcio da parte di Regioni come Puglia, ma soprattutto Veneto e Lombardia, che, mentre chiedevano maggiore autonomia con un *referendum*, mettevano a repentaglio quella che già avevano. A quel punto, siglato l'accordo, tutto dipendeva da come il Governo avrebbe dato attuazione all'accordo stesso nel decreto ministeriale annunciato per fine ottobre. la legge di bilancio 2016, quella di due anni fa, prevedeva che l'accordo Stato-Regioni sarebbe stato attuato con un decreto ministeriale, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari: un calvario, se il Ministro avesse forzato il testo contro le Regioni, dando adito a un'interpretazione più restrittiva; diversamente, rispettando le leggi regionali, si sarebbe esposto ad azioni da parte delle *lobby*, che prevedibilmente avrebbero preteso una diversa interpretazione di quell'accordo. Eravamo tutti in *suspense* ad attendere questo decreto, ma le vere intenzioni di Baretta erano puntualmente affiorate, con malcelata soddisfazione, subito dopo la firma dell'accordo: «Ora le Regioni non potranno più chiudere punti gioco» ha detto «ma solo decidere dove collocare quelli previsti». Ed ecco che, al posto del decreto, arriva la legge di bilancio; l'articolo 90 chiarisce definitivamente da che parte sta il Governo: lo confermano le velate minacce rilasciate pochi giorni fa di imputare alle Regioni un danno erariale qualora non depotenziassero le norme anti azzardo. Il danno erariale vale per le Regioni e non vale quando un Governo assegna una gara miliardaria *brevi manu*. perché non è arrivato il decreto? Perché, appunto, si trovava tra due fuochi e poi per un altro aspetto, molto più concreto. L'accordo stipulato il 7 settembre conteneva una lunga serie di previsioni, tra le quali alcune senz'altro virtuose e sgradite alle concessionarie; con questo articolo, il Governo lascia cadere nel vuoto le belle promesse e sul resto cerca di scaricare la palla alle Regioni. E, poiché la scadenza delle concessioni incombeva, ha cercato di divincolarsi dalla matassa che ha creato: creato: le convenzioni non si rinnovano finché le Regioni non si adeguano, ma nel frattempo i concessionari possono continuare a lavorare indisturbati, pagando un obolo. Dopo mesi e mesi di ben altri proclami, sul voler tutelare la salute, sull'aver compreso gli errori fatti in questi lunghi anni, di continui favori alle *lobby*, di continua liberalizzazione ed espansione di un mercato che ha raggiunto i 96 miliardi di euro, dopo le belle dichiarazioni sul voler

Il Sottosegretario dovrebbe prenderne atto e il Governo, che ha presentato in questo disegno di legge una norma tanto sconcia, dovrebbe fare altrettanto.

da una Nota di aggiornamento che ha ulteriormente scostato il cosiddetto obiettivo a medio termine, il che significa in parole povere maggiore *deficit*; è stato connotato da circa 16 miliardi per la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (per (per non aumentare l'IVA abbiamo dovuto impegnare tutte queste risorse) e, nel corso del dibattito, da una lettera dell'Unione europea che ci mette

3,5 miliardi di euro. Non sto parlando di polemiche, ma di lettere ufficiali; il che significa che un'attenzione rigorosa avrebbe dovuto essere esercitata

tutte o quasi dedicate alla spesa corrente e sempre in aumento della spesa corrente stessa. Questo, nonostante fosse già stato segnalato nel Documento di economia e finanza che la spesa corrente era aumentata di 2,5 miliardi,

statizzazione è una parola poco usata, desueta, che significa statalizzazione. Non abbiamo dato a questo nostro intendimento nemmeno la dignità

così irrigidendolo e ponendo le premesse per chi verrà dopo di trovarsi una situazione di finanza pubblica ancora più deteriorata. Infine,

che riguardano molti miliardi di euro), il Governo aveva dinanzi a sé una scelta: non usare ulteriori risorse per tentare il risanamento del bilancio o scommettere di usare risorse che abbiano una funzione

forse per il *superticket* durerà qualche giorno di utilizzo. È, quindi, una misura totalmente inefficace. Per la questione *bonus* bebè - uso il termine giornalistico - cioè per l'aiuto alle famiglie di minor reddito

sgranato questa manovra, rendendola così inefficiente. E allora, non abbiamo posto rimedio ai guai strutturali, che già sì profilano all'orizzonte, secondo quanto ci dice l'Unione europea, e alle risorse che disponevamo non abbiamo dato nessun indirizzo anticiclico anticiclico e, quindi, capace di aiutare lo sviluppo. Abbiamo fatto una cosa tutta sgranocchiata. Di contro, abbiamo certamente aumentato la la spesa pubblica con una serie di stabilizzazioni, statizzazioni o statalizzazioni, che dir si voglia. Signor Presidente, attenzione perché ciò significa dimenticare un concetto che - a mio avviso - è l'unico necessario reintrodurre in Italia perché si traduce, in termini culturali, in merito e, in termini economici, in produttività, che sono le uniche due cose di cui l'Italia necessita. Quando si fanno provvedimenti generalizzati il merito non c'entra e, anzi, viene penalizzato. Così questa legge di bilancio merita il nostro voto contrario e speriamo che sia l'ultima non della storia d'Italia, perché ci sarà quella del prossimo anno, ma l'ultima di questo Governo di sinistra.

Presidente, colleghi senatori, colleghi del Governo, la legge di bilancio stabilisce le priorità di un Esecutivo, di una maggioranza e di una forza politica rispetto alle spese del proprio Paese. Il testo che oggi discutiamo in questa Aula non smentisce questo assunto. È, infatti, lo specchio di un Governo e di una maggioranza che non hanno più una visione. alcune questioni di metodo, innanzitutto. L'esame in Commissione bilancio si è svolto nel *caos* più totale. In modo a dir poco grossolano sono stati falcidiati emendamenti con la tagliola dell'inammissibilità, per poi veder ripescati questi emendamenti, magicamente, di volta in volta che le proposte apparivano funzionali alle esigenze della maggioranza. È stato chiesto ai Gruppi di segnalare gli emendamenti più rilevanti entro un termine stabilito, ma tra inserimenti fuori termine e sostituzioni *last minute*, in alcuni momenti a tutto sembrava di assistere fuorché a un dibattito ragionato

dalla soluzione di questi problemi vi è stato chi ha tratto un indiscutibile vantaggio, come qualche Gruppo parlamentare che, dietro minaccia di far mancare il proprio voto decisivo, ha potuto beneficiare di una legge di bilancio *à la carte*. Passiamo ai contenuti. Se dobbiamo valutare con oggettività, non si può dire che non vi sia nessuna misura condivisibile. Anzi, di qualche aspetto positivo di questa manovra potremmo, senza timore di smentite, rivendicare il merito. Il problema è che, anche quando si è intrapresa la giusta direzione, ci si è fermati a metà strada in nome di altre e assai discutibili priorità.

In realtà, per certi aspetti questa legge di bilancio è invece la legge del «Non vorrei, ma sono costretto e dunque mi limito al minimo

80 a 40 euro al mese. Nemmeno sufficienti a coprire la spesa per i pannolini. Per non parlare della cifra destinata al fondo per il sostegno di coloro che si prendono cura di un familiare disabile grave: 7 euro a ciascuno di questi cittadini. La senatrice Bignami ha fatto di questa battaglia quasi una missione di vita, e noi l'abbiamo appoggiata. Mi sembra evidente che in questa legislatura sarà impossibile incrementare quella cifra simbolica, ma quel che si può fare è inchiodare Governo e maggioranza alle loro responsabilità, innanzitutto davanti agli elettori. A proposito di responsabilità, permettetemi di spendere qualche parola sulla vicenda delle banche. Permettetemi di farlo dopo due anni di battaglie dentro e fuori il Parlamento; dopo aver costretto il Governo, grazie a una mozione promossa dal collega Augello e portata avanti insieme a tutti gli altri Gruppi politici, a porsi il problema dei risparmiatori truffati fin qui esclusi dalle misure risarcitoria; dopo aver impegnato l'Esecutivo ad adoperarsi, attraverso misure interdittive efficaci, affinché gli amministratori responsabili dei dissesti non continuino a far danni Presidente, colleghi, è stata un grande successo l'approvazione unanime di un ordine del giorno che recepiva queste battaglie. Abbiamo atteso pazienti che il Governo mantenesse la parola data in quest'Aula e riconfermata anche dal sottosegretario Baretta a bordo del treno in questo periodo più famoso della politica italiana. Grazie alla mediazione del ministro Finocchiaro e del presidente Tonini siamo riusciti a far riammettere il nostro emendamento e a far sì che rimanesse fino all'ultimo sul sul tavolo della trattativa. I relatori hanno infine riformulato una proposta, in seguito approvata, che risulta però incompleta oltre che insufficiente da un punto di vista dello stanziamento. Infatti, 25 milioni di euro l'anno per tre anni sono briciole

perché questo inizio possa avere un seguito, è necessario che, come abbiamo fatto fino ad oggi, si continui a porre il problema a ogni livello istituzionale, con ogni atto possibile e su ogni tavolo decisionale utile.

anche per gli immobili commerciali; una proposta condivisa e presentata da vari Gruppi che poteva rappresentare, se ben congegnata a beneficio sia del proprietario che dell'affittuario, uno strumento per alleggerire gli oneri di locazione degli artigiani di bottega e dei negozianti. caso non è stato ritenuto fosse una misura degna di entrare in questo testo. Questa legge di bilancio avrebbe potuto essere anche un'occasione per attenuare un po' il carico fiscale che soffoca cittadini e imprese, per cercare di intravedere soluzioni - almeno parziali - per le pensioni dei giovani, per il riconoscimento di un trattamento pensionistico minimo a coloro che nella vita - spesso per necessità - si sono dedicati interamente alla cura della famiglia e degli anziani. Avremmo potuto tracciare un un solco per il presente e soprattutto per il futuro. Invece, si è ritenuto che meritassero di essere stanziati più di tre milioni per l'ippodromo di Merano, e si è pensato che potessero essere esonerati dagli obblighi di *spending review* gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (i cosiddetti IRCSS) pubblici e privati, senza considerare che probabilmente per fare un gradito regalo di Natale a qualche imprenditore sanitario vicino alla politica (o dentro la politica) si metteranno in crisi i fondi sanitari delle Regioni, che saranno costrette a nuovi tagli di servizi e prestazioni. Si è reputato anche opportuno spendere oltre tre milioni per la creazione di nuovi enti parco,

hanno trovato posto misure quali la deroga al *jobs act* per gli *steward* assunti dalle società di calcio, le deroghe agli obblighi di certificazione antimafia imposti dal codice degli appalti, il mille proroghe, le manifestazioni carnevalesche, i poligoni di tiro, misure in materia di società sportive dilettantistiche, la nuova Agenzia italiana del meteo, il registro nazionale dei procuratori sportivi, l'apicoltura in aree montane, il Piano di azione ONU sulle donne, la pace e la sicurezza. L'elenco sarebbe ancora lungo ma ve lo risparmio, perché già da queste brevi considerazioni è chiaro il disegno che sottende a questa legge di bilancio: concedere a pochi, possibilmente amici, per togliere a tanti. È singolare notare fino a che punto la deriva di un Governo che avrebbe dovuto rappresentare la sinistra moderna e riformista di questo Paese si sia spinta indietro. Ma questo, colleghi, lo lasceremo valutare presto agli elettori, tramite il voto. Io credo che oggi, nonostante queste considerazioni,

che questa fiducia vi renda ancor meno certi di avere quella degli italiani la prossima primavera. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Federazione della libertà alla fiducia posta dal Governo sulla legge di bilancio.

Io vorrei ragionare solo su un punto, anche molto brevemente, perché non serve spendere tanto tempo per spiegare questo concetto. Questa è una manovra di diversi miliardi, la gran parte dei quali sono destinati al superamento delle clausole di salvaguardia di salvaguardia e chiude cinque anni che sono iniziati all'insegna della prosecuzione del Governo Monti, che come tutti sapranno e possono ricordare è stato un Governo di emergenza dovuto ad una crisi finanziaria e politica di particolare rilevanza, di cui è chiara la responsabilità, sia sul piano finanziario ed economico, sia sul piano della gestione politica. Quel Governo, un Governo di emergenza ha costretto gli italiani - in una situazione nella quale l'economia era tracollata ed eravamo sull'orlo del baratro finanziario definitivo

ha fatto seguito un risultato elettorale non chiaro: non c'è mai stato al Governo un centrosinistra omogeneo; non c'è mai stata al Governo di questo Paese una maggioranza che sia stata espressa in modo coerente dall'elettorato. È stata una maggioranza che si è fatta carico, di volta in volta, modificando anche la sua natura, grazie. che ha portato il Paese dal segno meno al segno più e che ha consentito, per esempio, il superamento delle clausole di salvaguardia sull'IVA. L'IVA è una tassa ignobile, perché è una tassa indiretta; è sul prodotto, non è quindi proporzionata alla condizione condizione sociale ed economica del cittadino. Non segue il criterio della progressività. È una di quelle imposte che si pone sul fronte del consumo, spesso sul consumo destinato a famiglie e a persone che non sono in condizioni di particolare vantaggio. tutte le imposte indirette sono più inique delle imposte dirette perché queste ultime seguono il criterio della proporzionalità, indirette non lo fanno e non seguono neppure la condizione di bisogno, quindi di esigenza di lavoro, di vita, delle persone. superato quella situazione di crisi e aver sterilizzato le norme di salvaguardia è un grande risultato un grande risultato di cui bisogna tener conto. Ecco perché, rispetto alla situazione data, alle condizioni superate, oggi lo sforzo fatto dal Governo, e in modo particolare dal Ministro dell'economia, per tenere i conti e riportarli in salute merita il nostro voto favorevole. Io penso che consegniamo l'Italia in una condizione meno peggiore di quella in cui l'abbiamo ricevuta.

in fase di dichiarazioni di voto. sul testo A, e cioè prima che fosse posta la questione di fiducia dal Governo. Adesso, rispetto al maxiemendamento del Governo, abbiamo due ulteriori problemi: il primo è che non arrivava la relazione tecnica, la Commissione bilancio è convocata per le ore dunque, anche rispetto alla valutazione sulla ammissibilità delle parti dell'emendamento ordinamentali e localistiche non abbiamo ancora un responso. Abbiamo iniziato le dichiarazioni di voto senza avere ancora un testo legittimato. Mi permetto di dire che su quel testo ci dovrà essere anche il suo personale parere ed eventualmente la convocazione della Giunta per il Regolamento. il testo presentato dal Governo, rispetto a quanto dichiarato, non è interamente sostitutivo e corrispondente al testo A uscito dalla Commissione bilancio, ma è stata fatta almeno una modifica significativa per quanto riguarda i lavori socialmente utili.

anzitutto ringraziare, anche a nome della collega Comaroli, il vice ministro Morando, il presidente della Commissione Tonini, che non vedo, i relatori e - soprattutto - gli Uffici, per la mole di lavoro svolto nelle tante sedute della Commissione quali - diciamolo - sono state poco produttive, visto che la maggioranza, abusando del senso di responsabilità delle opposizioni, è stata impegnatissima a mercanteggiare emendamenti, spesso litigando al proprio interno. Emblematica è stata l'ultima seduta, terminata alle ore 5 di mattina - quella del saccheggio - durante la quale sono stati approvate a raffica decine di marchette. Questa è l'ultima manovra finanziaria della legislatura ed è tempo di bilanci delle politiche di questa maggioranza, sempre più dilaniata da scontri interni. Le cose non vanno affatto bene per il nostro Paese, nonostante il contesto europeo e mondiale favorevole. Noi cresciamo poco e in misura molto minore rispetto agli altri Paesi europei. Anche il divario tra la nostra disoccupazione e la media dell'Unione europea aumenta. Il nostro debito a settembre è a livello stellare, con 2.284 miliardi di euro. Siamo in difficoltà, come confermato dai magri numeri del disegno di legge di bilancio, pari a 20,4 miliardi tre quarti dei quali sono impiegati per neutralizzare le clausole di salvaguardia introdotte dal Governo Monti per evitare, ma - lo sottolineo - solo per il 2018, un catastrofico aumento dell'IVA. rimane poco: pochi nuovi investimenti e poche le misure per la crescita, il contrasto alla povertà e il sostegno alle famiglie. La manovra è in *deficit,* visto che è coperta, per oltre il 50 per cento, da 11 miliardi di nuovo debito. Le cose non vanno bene e lo sanno bene i cittadini, al di là delle favolette raccontate da Gentiloni Silveri e Padoan. Lo sanno i 7,5 milioni di italiani in stato di deprivazione, di cui 4,5 in povertà assoluta. Lo sanno gli italiani che rinunciano alle cure, perché non hanno i soldi per medicine ed esami. Lo sanno i tanti precari e i disoccupati, soprattutto giovani, che non trovano lavoro perché sempre più attività economiche chiudono per la crisi. Lo sanno i tantissimi italiani - oltre 120.000 all'anno, in gran parte giovani diplomati e laureati - che non vedono prospettive in questo Paese e preferiscono emigrare all'estero, magari per fare i camerieri a Londra o Parigi. Sì, questa manovra è negativa e inefficace e non risolve i problemi reali del Paese. Anzitutto, rinviate alla Camera dei deputati tante questioni cruciali, come la riforma delle agenzie fiscali per problemi tecnici, ma soprattutto politici. Rinviate questioni importanti riguardanti gli enti territoriali, prolungando per loro l'incertezza. Penso alle Regioni ordinarie e ai Comuni, che sono sempre più in difficoltà e, soprattutto, alle Province, sempre più sull'orlo del *default* per l'irresponsabile riforma Delrio. Innalzate ancora la spesa, stabilizzando altro personale nel pubblico impiego, oppure dando incentivi a pioggia senza alcun criterio meritocratico. Così, mentre spendiamo 5 miliardi all'anno per accogliere clandestini, restano poche risorse per gli interventi pensionistici, il sostegno alla famiglia e i risparmiatori truffati, inezie per il comparto difesa e sicurezza (ai nostri uomini in divisa non pagate nemmeno gli straordinari). Evitate l'aumento dell'età pensionabile a meno di 15.000 persone appartenenti a categorie usuranti, - ancora per colpa della maledetta legge Fornero - dal 2019 innalzate a sessantasette anni l'età per la pensione di vecchiaia e condannate la gran parte dei lavoratori a sgobbare per altri cinque mesi in più.

dato che da sempre sostiene che la riforma Fornero, con l'innalzamento repentino, abbia già inglobato gli aumenti dell'età pensionabile. Abbiamo presentato emendamenti anche per ampliare le salvaguardie. Insomma, proposte per creare un'uscita flessibile dal lavoro e attenuare la rigidità della Fornero c'erano:

mentre Renzi, cara relatrice Zanoni - che non vedo in Aula - il quale è in perenne campagna elettorale, promette ancora gli 80 euro per le famiglie numerose (e ricordo che lo fa dal 2014): di fronte all'allarme natalità non fate nulla per colmare sul territorio la carenza di asili nido e inoltre dimezzate il *bonus* bebè, prevedendolo non più triennale, ma solo annuale, con 40 euro al mese,

previsto per le misure di sostegno alle famiglie. Insomma, è il classico gioco delle tre carte. Continuate poi a beffarvi dei risparmiatori rovinati dai *crack* delle banche: per salvare il Monte dei Paschi di Siena, la banca del Partito Democratico, in passato avete messo diversi miliardi di soldi pubblici; per centinaia di migliaia di cittadini truffati vi limitate invece ad istituire un fondo di ristoro con soli 50 milioni in due anni, con la beffa però che i cittadini che devono dimostrare di essere stati raggirati con una sentenza passata in giudicato dovranno pagare avvocati e aspettare anni, per ottenere - forse - un ristoro che potrebbe risultare irrisorio; e allora molti rinunceranno. Avete anche ignorato e tradito le aspettative delle attività economiche, soprattutto delle piccole e medie imprese. Avete bocciato la cedolare secca per affitti di negozi e studi; avete cambiato le regole del gioco, rinviando di un anno l'entrata in vigore dell'imposta sul reddito Questo comporterà la mancata riduzione della pressione fiscale di 2 miliardi di euro, un danno enorme per 250.000 imprese che avevano già programmato la propria attività per il 2018. Avete impedito il riporto delle perdite per le imprese che applicano un nuovo regime di cassa, una grave penalizzazione per 2 milioni di imprese.

Mentre il Paese versa in enorme difficoltà, vedo tante facce sorridenti tra i colleghi di maggioranza e anche tra qualcuno che fa pseudo-opposizione: lo siete di più per quanto avete portato a casa per voi stessi che per il bene comune. Contentini, molte marchette e poche azioni strutturali ci sono in questa manovra. Non oso pensare cosa sarebbe successo se la *web tax* introdotta avesse portato gettito già a partire dal 2018: altro che assalto alla diligenza! Ribadisco tutto ciò succede mentre sprecate 5 miliardi all'anno per mantenere 200.000 clandestini, sedicenti profughi, che non scappano da guerre e si fanno beffa di noi. Molti di loro spacciano droga ai nostri figli, mentre altri sono dediti al traffico di prostitute: vengono beccati dalle nostre Forze dell'ordine e denunciati, ma, invece di essere espulsi, come in un Paese serio dovrebbe accadere, continuano a scorrazzare sul territorio. Mi avvio alle conclusioni. A questo punto, non bisogna perdere altro tempo per staccare la spina a questa maggioranza inaffidabile. Per altro, la lettera dell'Europa prefigura la necessità, a breve, di una manovra correttiva di tre, quattro o forse cinque miliardi, a causa dei conti pubblici non in ordine, per responsabilità della politica di Renzi, basata non su interventi strutturali, ma sui *bonus* e sull'aumento del debito. Lascerete un Paese con le macerie, come quelle presenti nelle zone terremotate del Centro Italia, e con le voragini nei conti pubblici. Questa è la vostra eredità fallimentare. Pochi italiani

per assecondare i tempi voluti dal Governo sul disegno di legge di bilancio. Non abbiamo ancora l'emendamento approvato dalla Commissione. La Commissione, forse, si sta riunendo in questo momento. Non so ancora se sia arrivata la relazione tecnica, non so quale giudizio di ammissibilità sia stato dato da quelle parti. Allora, vede signor Presidente, noi possiamo sostenere quello che vogliamo qui dentro ma se non abbiamo almeno il rispetto delle regole, diventa vuoto anche ogni parlare.

non come quello che abbiamo visto la scorsa notte, con un testo mancante di commi, non come quello che abbiamo visto in altre occasioni, con numeri sballati laddove è in ballo il destino di tante persone, aziende e famiglie. Ebbene, una sospensione dei lavori al fine di dar modo alla Commissione bilancio di completare il suo *iter* e, dopo, di valutare nel merito queste

Regolamento parlamentare che ha rango paracostituzionale. Stiamo dicendo che sono le regole di ingaggio o di collaborazione leale all'interno di quest'Aula. Non possiamo trattarle come un decreto-legge imposto con tempi forzati e con una mancanza di rispetto reciproco.

Signor Presidente, il vice ministro Morando ci ha ricordato i tre pilastri fondamentali della manovra: la sterilizzazione degli aumenti dell'IVA e delle accise, il rafforzamento delle detrazioni per gli investimenti privati, la decontribuzione per l'occupazione dei giovani. Su questo impianto ci sarebbe, secondo il vice Ministro, addirittura l'accordo di tutti. L'Ironia del Vice Ministro è però totalmente fuori luogo. I tre pilastri di cui parla sono effettivamente legati e dirò qualcosa su ciascuno di essi. È vero che tre quarti della manovra sono necessari per neutralizzare aumenti di IVA e di accise, decisi in larghissima parte con la legge di bilancio per il 2015, cioè con il primo Governo Renzi, Renzi, per finanziare misure specialmente di contribuzione e, in parte, di sostegno agli investimenti non coperte all'epoca. Si è trattato cioè di prenotazione di risorse dalle future leggi di bilancio, di cui oggi paghiamo il conto salato e lo pagheranno negli anni a venire i prossimi Governi, perché restano più di 12 miliardi per il 2019 e tra i 19 e i 20 miliardi negli anni successivi. Ora sterilizzare le cosiddette clausole di salvaguardia è un dato, un fatto dovuto, ma non rende la manovra espansiva, diversamente da quanto è stato sostenuto in quest'Assemblea. Significa solo evitare che sia molto depressiva. Un risultato anche questo, ma sicuramente molto poco esaltante. Tutto bene se avessimo avuto dalle misure finanziate in disavanzo gli effetti sperati; così non è però stato, né per quanto riguarda gli investimenti né per quanto riguarda il lavoro.

Qualcosa è stato fatto, viene riproposto nel settore privato, ma il tema che noi poniamo da tempo, con forza, è quello degli investimenti pubblici. Ora, la parola investimenti pubblici nella replica del vice ministro Morando non è nominata. Infatti gli investimenti pubblici sono passati dai 54 miliardi del 2009 ai 36 miliardi del 2016, con un calo del 35 per cento. Sono attualmente poco più del 2 per cento del PIL, poco più di quel che è strettamente necessario per gli ammortamenti delle strutture esistenti.

Noi sappiamo anche dagli osservatori internazionali, dal Fondo monetario internazionale per citarne uno, che gli investimenti pubblici hanno un moltiplicatore superiore al 2; ciò significa un impatto sulla possibile crescita economica molto forte, mentre gli strumenti cui facciamo ricorso a piene mani, cioè i trasferimenti e le detassazioni, hanno un impatto solo dello 0,7-0,8 per cento. La nostra è quindi una visione radicalmente diversa. Gli investimenti pubblici trascinano quelli privati; si pensi agli investimenti in infrastrutture, ricerca e sviluppo, nelle *utility*, nella protezione del territorio. La mancata messa in sicurezza del territorio non solo ha l'effetto di far perdere uno sviluppo significativo anche dal punto di vista della sua connotazione a favore dell'ambiente, ma ricordo che espone che espone a frane, valanghe e alluvioni che offendono la vita, la salute, la fiducia nel futuro, mettendo a rischio la coesione sociale dei territori e della cittadinanza. Per questo abbiamo avanzato proposte significative di rilancio degli investimenti pubblici, con un piano ambientale ad amplissimo raggio attraverso la riscrittura integrale, ad esempio, dell'articolo 95, con un emendamento che non credo possa essere sfuggito all'attenzione del vice ministro Morando che ha espresso un convinto convinto parere negativo.

Abbiamo visto invece degli incentivi, come ad esempio la diminuzione dell'IRES sui profitti delle grandi società, che non ha alcun ritorno, neanche dal punto di vista economico: si limita ad aumentare gli utili delle grandi società, delle grandi società, mentre invece alle piccole imprese nella legge di bilancio si fa una brutta sorpresa, cioè si pospone di un anno l'entrata in vigore dell'IRI, con un costo che si avvicina ai 2 miliardi di euro. È una piccola discriminazione ai danni delle piccole imprese. Parliamo adesso di lavoro di lavoro e qui le note sono molto dolenti. Ci vengono sempre ricordati - è stato fatto anche in questa Aula - i 900.000 posti di lavoro creati dalle decontribuzioni, non dal *jobs act*, che non c'entra niente, grazie ai quali abbiamo recuperato - ed è vero - il numero dei posti di lavoro persi con la crisi. però lavori a mezzo tempo, ad orario ridotto. Se noi non ragioniamo in termini di teste, di numero di lavoratori, ma di ULA, cioè unità di lavoro a tempo pieno equivalente quindi calcoliamo due *part-time* a mezzo tempo come un lavoratore - allora vediamo che il confronto con il 2008 è impietoso e lo dice l'ISTAT e non Maria Cecilia Guerra: siamo sotto di più di 1 milione di posti di lavoro a tempo pieno equivalente.

a tempo, a termine. Per questo abbiamo chiesto di intervenire su questo fenomeno reintroducendo le causali: niente da fare. Quanto al *part-time* si stima che 2,6 milioni di *part-time* siano involontari, ma sono spesso anche finti. Abbiamo chiesto più rigore nel controllo sui *part-time* finti e ci è stato risposto di no. Siccome anche noi consideriamo che il tema del lavoro dei giovani sia fondamentale, abbiamo voluto introdurre delle sanzioni per i falsi *stage*, quelli che non hanno contenuto formativo e che vengono utilizzati in sostituzione di lavoratori in malattia

Il tema è molto serio perché succedono cose veramente gravi che ci fanno capire la drammaticità della condizione dei lavoratori. Ricordo solo che ieri, con un SMS dalla FCA, l'ex Fiat di Cassino, sono stati licenziati 530 dipendenti interinali; ripeto, con un SMS*.*

è stata introdotta una deroga persino al lavoro intermittente. Non basta avere 18.000 tipologie di contratto, no; quelle che ci sono, nel caso dello sport, devono avere delle deroga per rendere ancora più facile e meno tutelato il loro utilizzo. Già la manovra, peraltro, per le società sportive è *for profit*: prevede non solo delle agevolazioni fiscali immotivate, visto che sono società che fanno profitti, ma prevede anche che, fino a 10.000 euro, possano assumere senza che ci siano imposte e, soprattutto, senza che ci siano contributi. Noi avevamo presentato un emendamento soppressivo di queste cose che consideriamo indecenti, ma il vice ministro Morando non li ha visti

negli effetti, sono frammentati nella platea, sono temporanei, non intervengono strutturalmente sui problemi. Faccio l'esempio del *bonus* bebè.

Se non si fanno gli asili e non si approvano gli emendamenti di altri, che sostenevano i servizi per l'infanzia, questo è contro la maternità. Se una lavoratrice all'Ikea prova a implorare che vengano adattati i tempi di lavoro perché è sola e ha due figli, di cui uno disabile, e viene licenziata questo è contro la maternità: altro che *bonus* bebè.

Ma questo succederà anche per i *caregiver*? È successo già per l'inserimento dei disabili. Attenzione: sono *spot* e durano lo spazio di un momento. Avete tradotto in *spot* anche il *superticket*, che è la nostra proposta da tempo. Questa cifra, che avete introdotto, sarà data alle Regioni perché ne facciano qualcosa di non ancora ben definito. Non avete capito che qui il problema non è dare un po' di soldi (che è sempre utile) ai più poveri; i più poveri già accedono al servizio sanitario. Il problema è che quel servizio sanitario deve essere universale; e se noi continuiamo, attraverso il *superticket*, a sbattere fuori dal servizio sanitario non i poveri, ma i ceti medi, quel servizio lì, che rimane solo per i poveri, si dequalifica.

mentre invece è passata una interpretazione autentica sui rigassificatori che fa veramente insospettire. Avete detto di no a un miliardo di altre proposte. Ne cito solo alcune perché il tempo è scaduto: la nona salvaguardia coperta dai soldi delle precedenti salvaguardie; la maternità, giustamente introdotta per le atlete ma non, ad esempio, per le allenatrici: ma perché? Non avete tenuto conto di una giusta osservazione: non possiamo calcolare la gravosità del lavoro dei braccianti agricoli con riferimento all'anno visto che lavorano a giornate. Tutte cose ragionevoli. Ma erano nostre; erano di Articolo 1-MDP e di Sinistra Italiana insieme a noi e non le avete accettate. Non vi siete occupati del tema dell'assegno sociale, che è una misura assistenziale e non può essere legata all'età contributiva, nonché di opzione donna, che abbiamo riproposto con forza. Poi, sono arrivate le mance e poi i milleproroghe e su quello avete dato ragione solo a chi ha "santi in Paradiso", cioè a chi ha un parlamentare forte della maggioranza. Quindi, solo alcuni territori hanno goduto di qualcosa, in modo casuale. E quanti parlamentari sono venuti solo a presidiare la loro mancia? Per i milleproroghe, poi, vi siete disinteressati di un tema importante che riguarda ventimila tra carrozzieri e gommisti che, per una proroga mancata, rischiano di non poter esercitare il loro mestiere dal 5 gennaio 2018, solo perché le Regioni in cui abitano sono state inadempienti nel fare i corsi di formazione necessari. Chiudo per dire che per tutte queste ragioni che riguardano l'impianto - vice ministro Morando che non ci sei - della manovra originaria, il metodo e il merito degli emendamenti, quello che c'è nella manovra e soprattutto quello che non c'è, il Gruppo Articolo 1-MDP voterà contro la fiducia richiesta dal Governo.

palesando le proprie idee, i propri convincimenti e le proprie legittime priorità, finanche nel nome del proprio Gruppo di appartenenza, si è limitato a snocciolare tutta una serie di nomi e sigle di aziende in crisi occupazionale, dopo aver votato aprioristicamente contro quelle proposte emendative a sostegno sostegno di un ricambio generazionale nel mondo del lavoro e a favore di alcuni ben determinati processi previdenziali. E pensare che ritenevo che queste fossero tematiche di sinistra! Ebbene, nel corso dei lavori in Commissione bilancio,

Aumentando il limite minimo dell'età pensionabile, non già per aziende o settori specifici, ma per tutte le società private con più di quindici dipendenti, abbiamo ottenuto un enorme successo nell'ottica di un ricambio generazionale sotto il profilo occupazionale; senza che lo Stato debba investire un solo euro, perché i costi di questa misura sono totalmente a carico delle aziende. Questa è stata certamente una significativa differenza tra chi in questi banchi si preoccupa esclusivamente delle chiacchiere e di comicità e chi, invece, pur esaltando, come già evidenziato, l'importanza e il significato del dibattito nelle Aule parlamentari, fa poi di tutto per passare dalle dalle parole ai fatti. Tradotto: le chiacchiere stanno a zero, perché quello che conta sono i fatti ed è innegabile l'eccezionale risultato ottenuto con l'approvazione dell'emendamento in questione a nostra firma, che creerà, nel prossimo triennio, circa 10.000 nuovi posti di

il post-pensionamento di quei medici che non fanno più i medici. Ci sono, infatti, circa 2.000 medici in Italia imboscati in attività amministrative, che sono fuori ruolo da oltre tre anni, che hanno infermità

i reparti e, quindi, ridurre i rischi della malasanità. Ovviamente il ministro Poletti non è riuscito a capire questa nostra proposta e noi riteniamo che abbia sbagliato; ciò non toglie che l'abbiamo fatta. Tuttavia un grosso risultato siamo riusciti a portarlo a casa. Passando invece al merito del testo sottoposto dal Governo al vaglio della Commissione, va detto che esso già conteneva misure improntate alla crescita e ritengo che nel complesso sia stato fatto un buon lavoro per migliorarlo ulteriormente, anche con gli oltre 150 emendamenti approvati,

Si va dagli incentivi per il lavoro, agli interventi in favore della famiglia e delle fasce più deboli della società, con un incremento dei fondi destinati alla lotta alla povertà. Essere riusciti a introdurre queste misure di grande impatto, specialmente sotto il profilo sociale, senza aumentare l'IVA o introdurre nuove tasse, è certamente un primo risultato importante che va riconosciuto all'Esecutivo. Anzi, una tassa è stata introdotta: la *web tax*.

dal suolo italico deve essere tassato, al 6 per cento. Credo che abbiamo fatto un gran lavoro, che nessuno aveva fatto prima. Un risultato tanto più soddisfacente, tenendo conto che si è, allo stesso tempo, riusciti a inserire anche parte di quelle misure a favore del Mezzogiorno che erano indispensabili già da tempo, sebbene sotto questo aspetto ci sia ancora molto da fare. Trovano il giusto spazio anche il pacchetto a favore delle imprese in tema di ammortamento e quello a sostegno degli investimenti pubblici, soprattutto per quanto riguarda gli enti locali con gli aumentati margini di spesa garantiti ai Comuni che potranno così impegnarsi anche per la riqualificazione delle periferie. Il tutto riuscendo anche a riconfermare gli *ecobonus*. Circa quanto invece introdotto al Senato, il nostro contributo è stato indispensabile per porre rimedio a quelle che sono, a nostro avviso, alcune dimenticanze del Governo, che abbiamo sanato proponendo interventi mirati in settori inizialmente completamente ignorati in questo disegno di legge di bilancio e non solo. Uno su tutti è il caso Ischia che, se non fosse stato per il nostro interessamento e per i nostri senatori campani, avrebbe rischiato di diventare un territorio di serie B rispetto a tutte le altre aree d'Italia colpite da calamità naturali, dai terremoti agli incendi, passando per le alluvioni, negli ultimi anni. È stato un lungo e costante lavorio che ha prodotto i suoi primi frutti già con il decreto-legge fiscale, recentemente licenziato dal Senato e che avendo luogo in questo momento la votazione sulla fiducia posta dal Governo. In quel provvedimento, infatti, si stanziavano ulteriori finanziamenti a sostegno delle popolazioni e degli enti dei territori interessati da eventi naturali straordinari e scandalosamente nulla si prevedeva per la ricostruzione e il rilancio di Ischia. Cosa ancora peggiore, e lo dico con sincero rammarico, alla distrazione del Governo in quella circostanza si era aggiunta quella di tutti gli altri senatori, essendo state quelle del Gruppo ALA non solo le uniche norme approvate per Ischia, ma addirittura le uniche presentate al decreto fiscale. Dopo l'istituzione di un fondo *ad hoc* per la ricostruzione, gli sgravi fiscali e tributari, la sospensione dell'IMU e le misure finalizzate alla ripresa economica di un'isola a vocazione quasi esclusivamente turistica inseriti nel precedente provvedimento,

È un successo di cui andiamo fieri e di cui l'intera Assemblea dovrebbe felicitarsi, perché abbiamo sanato quella che rischiava di porsi come un'ingiustificata ma soprattutto ingiustificabile ingiustizia Ho visto anche che questo emendamento è stato votato all'unanimità dalla Commissione, ma perché c'eravamo noi a permettervi di approvarlo. Abbiamo poi immaginato altre importanti previsioni, come gli interventi a sostegno delle Autorità di bacino da Nord a Sud della Penisola, al fine di ridimensionare il forte rischio Il nostro impegno si è però concentrato anche su tematiche specifiche che necessitano da tempo di risposte concrete, come la disciplina contrattuale degli *steward* negli stadi, rispetto alla quale abbiamo determinato un significativo passo avanti, considerando che allo stato

definendo ufficialmente in tal modo una figura professionale che finora non godeva di uno specifico inquadramento normativo. Orbene, alla luce di quanto detto, sento di poter affermare con certezza, mentre questa legislatura travagliata sta volgendo al termine, che abbiamo contribuito in maniera determinante a questo disegno di legge del finanziamento per 160 milioni del quadrilatero delle Marche e dell'Umbria.

il Gruppo per le Autonomie ha sostenuto in questa legislatura i Governi Letta, Renzi e Gentiloni Silveri. Lo abbiamo fatto sulla base di un patto politico e programmatico i cui esiti sono stati importanti anche per il Paese attraverso una costante e fondamentale azione di riforme politiche sostenibili di risanamento e la stabilizzazione dei conti pubblici. L'Italia - di questo si deve dare atto

stata una mirata e oculata politica fiscale come il superammortamento e la proroga dei *bonus* energetici per le ristrutturazioni. L'Italia è così sulla buona strada, anche se molto deve essere ancora fatto per eliminare il *gap* che registriamo rispetto alla media europea in ordine alla crescita del PIL. Siamo consapevoli che sia un obiettivo non facile, soprattutto in ragione dell'enorme debito pubblico accumulato che pesa come un macigno sull'economia reale e sulle risorse della finanza pubblica. Proprio per questo le riforme e i progressi fatti negli ultimi anni sono apprezzabili. Il punto di partenza e le condizioni politiche dell'Italia sono, infatti, molti più difficili rispetto ad altri Paesi europei. Per noi rappresentanti delle Autonomie speciali si chiude ora una stagione particolarmente positiva dopo gli anni bui del Governo Monti, che aveva minato la base e le fondamenta delle autonomie stesse. In questi quattro anni però abbiamo ripristinato tante cose che all'epoca sono state messe in forse, modificando ben quattro volte lo Statuto del

e ben tre volte con la procedura accelerata, ossia con la cosiddetta legge pattizia, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto. Questa via è praticamente tracciata anche per le trattative del Veneto e della e della Lombardia; lo stesso modello dovrebbe funzionare anche per loro. Mai nella storia, dal 1948 in poi, è successo

Con la legge di stabilità del 2014 abbiamo ottenuto la competenza primaria per i tributi locali e per la finanza locale. Ciò ha consentito al legislatore provinciale di sostituire l'IMU con l'imposta provinciale sugli immobili, un sistema, a nostro parere, molto più equo rispetto a quello vigente nel resto del Paese perché non prevede l'esenzione totale sulla prima casa e, quindi, anche dei villini o degli appartamenti di lusso, ma solo per i primi 100 metri quadrati (mentre sul resto si paga). Si evita così una progressione inversa che permette di risparmiare di più a chi è più ricco. Con il maggiore gettito derivante da questa esenzione parziale sulla prima casa abbiamo abbassato l'imposta sui capannoni e gli alberghi, favorendo così il settore produttivo e i servizi. Penso che anche per questo motivo la crescita nelle nostre Province è superiore alla media nazionale. Siamo orgogliosi di questo provvedimento e anche della fiducia che il Parlamento nazionale e il Governo ci hanno dato, perché crediamo di aver introdotto una norma virtuosa che è generalmente accettata dai cittadini e molto apprezzata dalle imprese, anche se questa volta c'è un trattamento inverso: mentre a livello nazionale non si paga per la prima casa, in Provincia di Bolzano si paga per la prima casa se ha più di 100 metri quadrati. Un'ulteriore importante modifica dello Statuto riguarda l'accordo finanziario introdotto con la legge di stabilità del 2015: il cosiddetto patto di sicurezza. Anche questo va detto una volta tanto in quest'Aula: si tratta di un accordo con il quale abbiamo accettato praticamente tutti i tagli fatti dai precedenti Governi, versando ciascuna Provincia

la certezza che non ci saranno ulteriori tagli e che possiamo fare una programmazione seria dei lavori e del nostro bilancio. Si può quindi dire che non è vero che le Province di Trento e Bolzano hanno un residuo fiscale molto minore rispetto alla Lombardia. La Provincia autonoma di Bolzano, ad esempio, è più o meno ai livelli del Lazio: oltre 2.000 euro per abitante va

l'opposto. Con la presente legge di bilancio si attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano anche un'altra modifica dello Statuto sulla competenza primaria sulle concessioni idroelettriche. Dal 1° gennaio 2018 le Province potranno disciplinare i collegi provinciali, i criteri e le regole di attribuzione di queste concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (una delle maggiori risorse delle nostre Province). si determinerà il completamento delle competenze provinciali in ambito energetico, iniziato nel lontano 2000 con la delega, a suo tempo fatta dal Governo D'Alema, delle funzioni amministrative nell'ambito delle concessioni idroelettriche. Non ci sono quindi oneri maggiori per la finanza pubblica, perché l'intero gettito dei canoni di concessione già oggi spetta alle due Province. Inoltre, siamo riusciti a sbloccare l'erogazione delle quote variabili spettanti da tantissimi anni, ma mai erogate

Concludendo, consentitemi, colleghi, una considerazione. Se il Governo spagnolo avesse avuto anche solo il 10 per cento della sensibilità del Governo italiano, oggi forse non si porrebbe la questione catalana. Ringraziamo in particolare il vice ministro Morando ma anche il ministro Finocchiaro per la loro particolare sensibilità

che sono proceduti i lavori, ma anche per il loro rispetto per il lavoro dei singoli parlamentari, esaminando uno per uno i tanti emendamenti sia di maggioranza che di opposizione. Ringraziamo anche il presidente Giorgio Tonini per la sua bravura e per il suo equilibrio nella conduzione dei difficili lavori in Commissione bilancio, e i due relatori Zanoni e Gualdani, che hanno contribuito a creare un clima molto positivo e costruttivo per i lavori in Commissione. Per queste ragioni, il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE esprimerà voto favorevole alla fiducia posta dal Governo.

Lo faccio, signor Presidente, soprattutto perché oggi ho sentito, ancora una volta, portare dati entusiastici e rivendicazioni di successi,

un'impostazione che si è contraddistinta essenzialmente in quasi tutte le manovre di bilancio per una sorta di politica di *bonus* da una parte e di incentivi dall'altra, sempre con la caratteristica di essere non finalizzati ma a pioggia. Solo di *bonus* abbiamo calcolato in questi anni un ammontare di 62 miliardi

a pioggia, sarebbe stato necessario e poteva essere molto più produttivo concentrare invece questi 62 miliardi di euro in piani di investimento che sono il vero punto

su cui è possibile operare, a nostro avviso - di investimenti pubblici; che potesse davvero permettere in qualche modo di favorire l'occupazione e di sostenere importanti piccole e medie opere, investendo sul territorio, nelle ristrutturazioni edilizie, nella cura contro il dissesto idrogeologico, nei trasporti pubblici; un piano di investimenti che, come si fa nei Paesi seri, potesse davvero permettere di darsi una scrollata e uscire dalla crisi.

su cui questa manovra è stata incentrata - tra l'altro dicendo falsità, ovvero che nessuno ha presentato piani alternativi, e ma su questo punto tornerò - conferma questa impostazione che noi riteniamo assolutamente sbagliata.

è evidente a tutti che questo è dovuto più che a fattori interni, a fattori esogeni; questo lo sanno tutti, basta vedere le analisi macroeconomiche. È evidente che questa piccola ripresa, questo avanzamento, è legata soprattutto al basso costo del denaro e delle materie prime. prime. Approfittare anche di questa contingenza più favorevole significava allora investire per consolidare e mettere gli assi fondamentali di questa ripresa economica; perché la ripresina, come è arrivata per fattori esogeni, se ne può riandare. Altra rivendicazione che continuate a fare:

Inoltre, continuate ostinatamente a pensare che attraverso il meccanismo della decontribuzione, questa volta per i giovani, si possa favorire l'occupazione giovanile, ma questo non accadrà, sarà ancora una volta una cosa molto vaga e non consolidata. Invece continuate con la

a vedere gli emendamenti per distribuire le mance, per favorire le nuove coalizioni e per consolidare e avere i voti di fiducia per guardare attentamente le proposte che abbiamo presentato.

per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio, per il trasporto pubblico, per la qualità della vita. Invece vi siete ostinatamente rifiutati di prendere in considerazione non solo la proposta più generale del piano investimenti, ma anche le proposte ancora più

Noi abbiamo presentato una proposta seria di eliminazione del *superticket* e una proposta seria sul problema della denatalità, perché siamo intervenuti con proposte adeguate che riguardavano, per esempio, il sostegno al lavoro delle donne abbiamo presentato proposte significative per quanto riguarda gli asili nido e la scuola dell'infanzia. Perché non basta avere quattro briciole per sostenere i bebè, quando poi non c'è niente per la scuola dell'infanzia, per il lavoro. Il motivo vero per le donne per cui non si fanno figli è che i giovani pensano di poter mettere su famiglia a quarant'anni, perché c'è il problema drammatico del lavoro dei giovani.

Quindi, avete poco da vantarvi dei risultati, perché è tutto fittizio. Noi continuiamo a essere comunque fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la crescita e ad avere il *record* dei giovani che non studiano, né lavorano (pari a quasi il 20 per cento). Questi sono i problemi. Abbiamo il problema della povertà e pensate voi, con queste piccole misure, di essere in grado di affrontare il dramma di 4,5 milioni di persone che sono in stato di povertà? Questi sono tutti temi che non avete voluto affrontare,

Questo sarebbe il piano ambientale. Questa sarebbe la strategia di decarbonizzazione che avete messo in atto: fare l'abbono per milioni e milioni di euro

Do la parola al presidente della Commissione bilancio, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.700. *(PD)*. Signor Presidente, la Commissione bilancio si è riunita, come da prassi ormai consolidata, per verificare i profili di copertura del maxiemendamento, nonché la sua corrispondenza al testo approvato dalla 5a Commissione in sede referente. Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè i profili di copertura, il testo di riferimento è anzitutto la relazione tecnica, che è positivamente verificata e bollinata dal Ragioniere generale dello Stato. In calce alla firma del Ragioniere si legge la seguente nota: «La relazione tecnica è verificata positivamente, a eccezione dei seguenti commi: commi da 107 a 110, in quanto comportano maggiori oneri non compensati, sottostimati nella previsione contenuta nel testo e a carattere strutturale crescente;

La 5a Commissione raccomanda quindi al Governo di adempiere a questa condizione posta dal Ragioniere generale dello Stato e di espungere questi commi dal testo. Trattandosi di commi che riguardano un argomento socialmente molto sensibile, cioè il tema dei lavoratori che sono stati esposti a lungo agli effetti negativi, talvolta letali, dell'amianto, la Commissione raccomanda al Governo, che naturalmente deve adesso espungerli, di riprendere l'argomento alla Camera. Ovviamente, poi, sarà la Camera dei deputati a decidere in piena autonomia, ma credo che il Senato possa raccomandare al Governo di riproporre la questione alla Camera, naturalmente di correggere i profili di copertura ma di mantenere alta l'attenzione su questa categoria di lavoratori particolarmente colpita particolarmente colpita dalle vicende della vita e del lavoro. Dal punto di vista, invece, della corrispondenza del testo del maxiemendamento al testo approvato dalla

al comma 316, che corrisponde al comma 3 dell'emendamento 49.0.8 (testo 2)

il comma 344 che corrisponde al comma 2 dell'emendamento 54.0.33 (testo 3). Siamo nell'argomento delle misure per gli LSU della scuola di Palermo. Qui è stato riformulato il comma 2 che, nel testo approvato dalla Commissione, effettivamente, forse con un eccesso di genericità, diceva: «Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni» per limite nostro evidentemente, non è stato definito da parte di chi deve essere pubblicato il bando. Il comma è riformulato nel maxiemendamento con la dizione: «Con decreto del Ministro dell'istruzione assenso del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, è definito apposito bando». La Commissione suggerisce, a sua volta, al Governo che forse sarebbe più opportuno dire «Ministero», posto che si tratta di un atto che forse può essere di tipo di tipo dirigenziale. Comunque, ci rimettiamo al Governo per risolvere questo problema, che evidentemente è relativo definizione compiuta di un testo, che peraltro è chiaro nei suoi intendimenti. Concludo, Presidente, con i ringraziamenti per quanti hanno lavorato in Commissione bilancio in questa maratona. È stato già fatto oggi dai relatori, quindi non mi ripeto. Io vorrei concentrarmi nel ringraziamento al personale della 5a Commissione *(Applausi)*

il presidente Tonini, da 107 a 110 e il comma 144. S'impegna contemporaneamente

In secondo luogo, il Governo riconosce senz'altro la mancata corrispondenza, al comma 316, tra il testo approvato in Commissione, che noi avevamo fermissima intenzione di rispettare, e il testo così come era nel

il riferimento al Ministero in tutte e tre i casi e non al Ministro. Direi che queste sono le osservazioni che sono state fatte, che il Governo accetta. Infine, signor Presidente, se lei è così gentile da seguirmi un attimo, si tratterebbe di eliminare dal testo un vero e proprio refuso.

provvede (…)». Nel caso di questi emendamenti abbiamo provveduto a fare una copertura su fondi, che è di tipo generale e contiene il riferimento ai commi, con il risultato che se lasciassimo questa dizione al comma al comma 206, esso, sia pure per una cifra bassissima, sarebbe coperto due volte. È una sovracopertura che sarebbe meglio eliminare,

«La Commissione propone, su proposta del senatore Arrigoni»,

visto che abbiamo ringraziato tutti, visto che abbiamo regalato prebende a tutti con gli emendamenti, almeno rispettare la parola data in Commissione con un senatore, che comunque si era impegnato. Le parole del senatore Tonini pesano e, di conseguenza, è giusto che le promesse vengano rispettate. TONINI *(PD)*. Le parole pesano come il senatore Tonini. Certo: è

Aggiungo allora, per completezza perché lo avevo dimenticato, che qualche senatore ha avuto da eccepire sulla contemporaneità della seduta della

valido su cui discutere e su cui dichiarare poi il voto. Sono ancora in attesa della valutazione della 1a Commissione, a meno che non la si voglia dare per implicita, sull'ammissibilità delle parti ordinamentali e su quelle localistiche inserite a piene mani dal Governo e dalla maggioranza di Governo durante tutto l'*iter* della manovra. Vorrei che il presidente Tonini esplicitasse questa considerazione, perché qui, nel Palazzo, le persone che lavorano con noi e che hanno esperienze delle passate legislature, mi dicono che non si è mai vista un'ammucchiata di interessi come in questa legislatura

o giù di lì per le vittime dell'amianto, rifiutando 80 milioni di euro che sarebbero derivati dall'abolizione dei vitalizi. Né l'una, né l'altra misura sono state inserite,

Per quanto riguarda poi le dichiarazioni, è chiaro che tutto ciò che è stato ritenuto non compatibile in relazione alle funzioni della Commissione è stato dichiarato; tutto il resto,

mi preme specificare che il Presidente della Commissione bilancio ha fatto un intervento esatto e corretto, mentre il Vice Ministro, nel

Alternativa Popolare è pronta a dare la propria fiducia al Governo, così come è stato chiesto. In tema di *bonus* bebè, voglio specificare ancora una volta che noi abbiamo fortemente apprezzato

Abbiamo assistito anche a vivaci interpretazioni. Così come ho avuto modo di richiedere ieri al Governo di precisare, proprio per evitare vivaci interpretazioni, dal momento che abbiamo ascoltato il capogruppo Santini in Commissione bilancio dichiarare che la Commissione aveva votato un determinato provvedimento, cioè la triennalità per le famiglie (quindi non solo un anno), io tengo qui a ribadire la conferma delle dichiarazioni del vice ministro Morando e che l'accordo, sia politico che strategico, sulla famiglia è stato rispettato dalle sue dichiarazioni. Proprio per queste interpretazioni vivaci, il Governo, se lo riterrà, interverrà alla Camera. Saremo attenti anche noi qui in Senato, proprio per il lavoro che verrà fatto alla Camera e per le scelte che saranno prese, soprattutto alla luce del fatto che spetterà proprio a quest'Aula e a questa Camera l'approvazione definitiva, ovvero la terza lettura. Voglio anche ribadire un convinto sì su determinati aspetti che riguardano, come dicevamo ieri, impresa, lavoro e famiglia. Per quanto riguarda la famiglia, il nostro impegno continua, oltre che sul *bonus*, su un riconoscimento delle detrazioni per i figli a carico, che spero la Camera riesca a portare a compimento. Sul tema delle imprese abbiamo fortemente apprezzato la volontà di creare la decontribuzione per i nuovi assunti nel Mezzogiorno. Le aziende che assumeranno giovani fino a trentacinque anni nel Mezzogiorno potranno beneficiare di questa decontribuzione. È un fatto molto importante e concreto, perché spesso siamo stati accusati di non intervenire al Sud e di trascurare il Sud. Una decontribuzione di questo tipo indubbiamente è un grande riconoscimento.

Il *superticket* viene destinato a soggetti più vulnerabili. Siamo assolutamente consapevoli che le risorse non potranno soddisfare tutte le esigenze: arriveremo fino a un certo punto. La Camera, lo ripeto, potrà anche apportare dei miglioramenti, ma per noi è importante avere ripristinato il principio che i più deboli, i più vulnerabili e anche i bambini possono beneficiare di un abbassamento del *ticket* rispetto agli altri cittadini.

Concludo ringraziando veramente, per la grande fatica e per il grande sforzo che è stato compiuto da parte di tutti, da parte del Governo, da parte dei componenti della Commissione bilancio, da parte dei relatori, del nostro relatore senatore Gualdani e della relatrice Zanoni.

Comunque senatrice Vicari, visto che il Governo si è pronunciato per impegnarsi per le vittime dell'amianto, ancora una volta è dimostrato che il bicameralismo è utile. Ne prendiamo atto.

Presidente, ho ascoltato nella discussione generale, nelle dichiarazioni di voto e nelle repliche dei relatori e del Governo così tanti ringraziamenti, così tanta autocelebrazione di quanto si è stati bravi. Vorrei anche ringraziare il vice ministro Morando, dal momento che si è così impegnato nell'approfondire 4.000 emendamenti: lo immagino alla ricerca del nostro emendamento sul reddito di cittadinanza, che questa mattina, dispiaciuto, mortificato, ci ha detto non essere riuscito a trovare. Ebbene, non è riuscito a trovarlo perché noi non lo abbiamo presentato, perché per cinque anni di seguito lo abbiamo fatto per sentirci dire sempre no, e perché è incardinato in Commissione lavoro e qualora il Governo volesse portarlo avanti, noi saremmo pronti. Ma, dal momento che, evidentemente, non vuole e dal momento che il Movimento 5 Stelle viene sempre accontentato pochissimo o quasi niente, avevamo avevamo deciso di puntare su un altro emendamento, che eravamo certi che il Partito Democratico avrebbe recepito, perché, di fatto, riprende un suo disegno di legge, a firma Richetti.

sull'andamento dei lavori, perché esso - lo dico per chi non ha assistito ai lavori - è stato piuttosto deprimente. Oltre al fatto che abbiamo il Governo sotto scacco di ALA, il Gruppo di Verdini, che l'ha costretto anche a cambiare parere su un emendamento ben specifico.

di essere denigrati, offesi da uno che è condannato in primo grado per il *crack* di una banca *(Applausi dal Gruppo M5S)*, da un nostalgico di un latitante - e sto parlando di Barani - e da un altro che è solo bravo a fare insulti sessisti e a dire che le donne devono girare ben

Signor Presidente, effettivamente, insieme a Barani e Verdini, quando ho parlato degli insulti sessisti, avevo dimenticato il senatore D'Anna; dal momento che non è stato nominato probabilmente si è offeso.

riservato un trattamento diverso; eravamo convinti che ci fosse più serietà, che sicuramente ci sarebbe stato un dialogo costruttivo, perché noi ci siamo messi lì e abbiamo proposto emendamenti di buonsenso, rispetto a un Governo che, comunque, è anche in scadenza. Ho sentito in quest'Aula parlare di crescita, di consegna di un Paese migliore. Allora vorrei ricordare al Governo, a quella diminuzione delle tasse che adesso vanno vantando, che si tratta di 15 miliardi per bloccare le clausole di salvaguardia, ma le clausole di salvaguardia, che - ricordiamo a chi ci ascolta da fuori - non sono altro che un aumento di IVA o di accise o comunque un aumento di tasse che sono poste in bilancio per coprire eventuali buchi, non le abbiamo inventate noi: sono di qualcuno e hanno un origine ben precisa. Le clausole di salvaguardia

Renzi poi le fa diventare esponenziali: 16, 19, 22 per cento, per tre anni. Poi cominciano una serie di cavilli, di false evasioni fiscali fatte di condoni fiscali, mentre sono andati a strozzare le nostre aziende, quelle che lavorano con Stato e che con lo *split payment* non hanno la liquidità per affrontare questo sistema che le strangola. E così loro fanno finta di fare la lotta all'evasione fiscale, le imprese e rimandano una valanga sempre più grande al Governo che verrà. E quando al ministro Padoan e all'Ufficio parlamentare di bilancio ho chiesto: secondo voi, dopo tutta la flessibilità ottenuta dell'Europa, sarà possibile non aumentare le tasse? No, non è possibile. Perché la crescita, che è stata assimilata grazie alle politiche di questo Governo, non sarà in grado di assorbirla. E parliamo di crescita. Qualche settimana fa ho partecipato a un incontro molto interessante, organizzato dal centro studi «Economia Reale» con il professor Baldassarri, il quale, con un'analisi controfattuale estremamente interessante che davvero propongo a tutti i parlamentari di analizzare e approfondire, ci ha detto, con i numeri, i dati e le tabelle, che se non ci fosse stata l'opera di Draghi del *quantitative easing*, fino al 2017 avremmo avuto sempre una crescita negativa. Noi siamo riusciti, rispetto al resto d'Europa, a frenare l'azione di Draghi con le politiche del Governo Renzi, Berlusconi e anche Gentiloni Silveri, perché sono tutti un'allegra compagnia, dove si sono scambiate una serie di mancette e sono stati accontentati tutti: persino la parrocchia di sotto

di bilancio sono andati a cambiare il codice civile per aiutare le cooperative e sono andati a derogare al codice degli appalti, approvato quest'anno, e al codice antimafia approvato quest'anno! Non sapete legiferare, perché poi andate in deroga e ALA).* È così. Il disegno di legge di bilancio è stata fatta di deroghe e del milleproroghe, che già non ci dovrebbe essere, ma lo avete infilato lì. Ma sì, tanto che fa, ce ne dobbiamo andare tutti a casa, al collegio elettorale.

quando è arrivata la Presidente della Commissione sanità che si è messa a battere i piedi come una bambina della scuola materna, perché voleva la prima firma da portarsi a casa

imbarazzante è stato vedere tutti i parlamentari, compreso adesso ancora Centinaio, rivendicare una prima firma del piccolo onorevole che vuole l'emendamentino da portarsi

i truffati dalle banche. Ma noi abbiamo votato favorevolmente perché quell'emendamento, quella scelta politica smentisce il segretario del Partito Democratico Renzi che, a Radio 105, ha detto che quelle persone sono degli speculatori.

caratterizzata da importanti interruzioni necessarie per tenere unita una maggioranza eterogenea. La legge di bilancio è stata gestita con modalità che oserei dire innovative e che, nel testo uscito dal dibattito in Commissione, non ha tenuto conto di alcune indicazione che veniva dalle forze di opposizione. A tutte queste evidenti scollature abbiamo voluto rispondere con tanto buonsenso, che poco è stato sottolineato in questa Aula per il grande rispetto che portiamo verso i cittadini. Tre sono i concetti chiave di questa legge di bilancio: pochi soldi, necessità di tenere cucita una maggioranza che ha difficoltà a trovare una linea comune di intenti e poche idee su come impegnare le scarse risorse. La strada stretta indicata dal ministro Padoan è il limite di questa legge di bilancio e noi la strada stretta l'abbiamo vista molto bene. Forza Italia ha puntato per questo su pochi e selezionati obiettivi: più aiuti alle nostre famiglie, sempre più stremate da questa crisi; maggiori interventi per la sicurezza e l'immigrazione; qualche misura per cercare di far ripartire il Paese come - per esempio - l'introduzione della cedolare secca per le attività commerciali. Qualcuno stamattina ha detto che non abbiamo presentato le nostre bandiere, come l'introduzione di una pensione minima più accettabile. Dopo quattro anni di leggi di bilancio in cui abbiamo presentato le nostre proposte, che non avete

La maggioranza - come ho già detto - non ha colto nessuno dei nostri temi. Ha inserito qualche nostra idea nella formazione dell'emendamento sul *bonus* bebè, ma senza cogliere l'essenza del problema: in un Paese dove il calo della natalità è inesorabile, la soluzione non sono gli 80 euro (che poi scenderanno a 40 dal 2019) assegnati a chi ha un ISEE molto basso. Inquadriamolo piuttosto come un *bonus* povertà, perché come molte delle misure proposte in questi anni sono servite solo a tamponare la crescita di situazioni di marginalità sociale. In questa legge di bilancio l'intervento sulle pensioni ha formulato una disposizione sui lavori usuranti che non è né giusta, né introduce princìpi di equità per gli anni a venire; ancor meno nei confronti delle nuove generazioni, da sempre tutelate a parole dai Governi Renzi e Gentiloni Silveri. Si inseriscono alcune categorie in modo molto parziale e se ne lasciano fuori altre che, magari, solo per la ripetitività del compito, che già di per sé produce produce usura, avrebbero avuto la priorità. La proposta sulle pensioni va - a nostro giudizio - nella direzione sbagliata. Ci sono voluti vent'anni per riuscire a unificare un sistema previdenziale nel quale ogni categoria aveva le sue regole e i suoi requisiti di età. Ed ora che finalmente abbiamo un sistema unico e universalistico, stiamo reintroducendo differenze tra lavoratori. L'unica soluzione - secondo noi - è inserire una serie di flessibilità in uscita. Oggi, la nostra sfiducia è non solo su questa legge di bilancio, ma è nel complesso dei provvedimenti adottati in questi anni dai Governi di sinistra. Aumentano i poveri e, anziché creare nuove ricchezze e favorire una crescita economica strutturale, si sono poste solo le condizioni per redistribuire la ricchezza esistente, rendendo necessari nuovi interventi per attenuare il crescente disagio sociale. Ormai l'effetto Francoforte è chiaro e ancora una volta bisogna ringraziare il presidente Berlusconi per avere trovato il consenso europeo su una figura di assoluto prestigio come Mario Draghi a guidare la Banca centrale europea. Le variabili esogene estremamente positive esplicano ora appieno i loro effetti sui nostri conti pubblici con una crescita stimata tra l'1,5 e l'1,6 per cento per quest'anno, ma in diminuzione all'1 per cento già dal 2018 e per gli anni a venire. Anche queste previsioni confermano la mancata spinta dell'azione riformista

Come ogni anno, l'attenzione sulla manovra di bilancio si è concentrata sugli interventi normativi contenuti nella prima parte, quella che tradizionalmente era la legge finanziaria e poi legge di stabilità. La seconda parte, quella che riguarda il bilancio dello Stato vero e proprio, sarà per il 2018 largamente a politiche invariate; una legge di bilancio da 860 miliardi, una prima parte che vale 20 miliardi e le modifiche introdotte dalla Commissione che valgono poco più di 600 milioni di euro. Quindi, per effetto delle modifiche apportate, È facile capire che questa manovra, esattamente come le precedenti, non cambierà lo stato complessivo dell'economia italiana. Rimangono un carico e una pressione fiscale opprimenti che si riducono solo in conseguenza della crescita del denominatore, il PIL, per le cause esogene di cui ormai troppo spesso parliamo tutti. Viene rinviata l'introduzione dell'IRI, una misura attesa soprattutto dai piccoli imprenditori, mentre permane una spesa pubblica che è largamente centralizzata e in larga parte improduttiva. Una parte preponderante del debito pubblico è appostata soprattutto a livello centrale e non negli enti territoriali. Eppure, ancora una volta c'è l'ennesimo sacrificio di 2 miliardi viene chiesto alle Regioni. Il problema della riduzione delle tasse non è al centro dell'agenda di questo Esecutivo, né lo è stato in quella dei precedenti Esecutivi Oggi, questo Governo non solo non riduce la pressione fiscale, ma la aumenta. Dei 21 miliardi di minori entrate, 19 sono utilizzati per la sterilizzazione delle clausole IVA del 2018 e il differimento dell'entrata in vigore dell'IRI sulle imprese, come ho detto qualche minuto fa. Dall'altra parte, ci sono più di 11 miliardi di entrate, che sono vere e proprie imposte o tasse. Cosa manca allora? Manca un autentico intervento strutturale sulle regole della nostra economia a partire dal sistema fiscale e dal sistema burocratico; un serio piano per dare un moltiplicatore agli investimenti pubblici. Ovviamente nulla viene fatto per estinguere i debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori di beni e servizi, mettendo in ginocchio tante, troppe aziende e tanti, troppi lavoratori. Le ragioni per cui non possiamo votare la fiducia a questa legge di bilancio, quindi, le rappresentiamo non solo noi oggi in quest'Aula, ma anche gli imprenditori abbandonati, i lavoratori autonomi oberati di tasse e burocrazia, i lavoratori dipendenti che godono di un mercato del lavoro non inclusivo. Tutti loro manifestano un dissenso verso l'azione di questo Esecutivo che è palpabile ogni giorno da chi vive tra la gente e con la gente. Per queste ragioni, Forza Italia oggi esprime il suo no a questa ennesima fiducia. Grazie. la legge di bilancio oggi in approvazione conclude gli interventi di politica economica sviluppatisi in modo articolato nel corso dell'intera legislatura e agisce dentro margini molto stretti, in quanto responsabilmente il Governo ha deciso di dedicare tre quarti dell'intervento alla disattivazione delle clausole di salvaguardia, per evitare di aumentare la pressione fiscale diretta e indiretta sulle famiglie e sulle imprese. La legge di bilancio, nella lettura del Senato, ha scelto di misurarsi in modo non riduttivo con i temi che riguardano le condizioni di vita delle famiglie e delle imprese, posti Grazie. pongono a tutti i Paesi un tema nuovo che riguarda il ritmo della crescita e le politiche di sostegno possibili in un contesto di vincoli di bilancio stringenti e di bassa inflazione. Di fronte a questo, sono stati posti interventi di sviluppo per quanto riguarda sia l'occupazione, sia gli investimenti. Inoltre, le trasformazioni sollevano anche il problema dell'avanzare dell'economia digitale, che pone la questione di come tracciare fiscalmente le attività economiche e come adeguare il capitale umano e gli investimenti a questi cambiamenti. Si sono date risposte importanti sull'occupazione giovanile, che è la più colpita in questo momento; sull'impegno a sostenere gli investimenti innovativi, sia nella quantità che nella qualità, e sul fatto di rafforzare il capitale umano dei nostri giovani con interventi specifici portati nella legge di bilancio. Inoltre, proprio qui al Senato si è introdotta la *web* *tax*, che rappresenta una prima risposta La seconda grande trasformazione è la crisi demografica, che pone da anni e porrà sempre di più in futuro molte domande sociali, a partire dal tema affrontato nei provvedimenti. Qui abbiamo visto in modo approfondito la questione previdenziale, disegnando una percorso che, nel necessario mantenimento dell'equilibrio della spesa complessiva previdenziale adesso e nel tempo, ha permesso però di aumentare la protezione sociale a 15 fasce di lavoratori che non potranno prolungare la loro permanenza al lavoro, introducendo altresì il tema di come differenziare, con dati scientifici, il calcolo dell'aspettativa di vita e il correlato incremento dell'età di accesso alla pensione sulla base di una decisione che verrà legata alla gravosità dei lavori. Questo è un elemento importante di riforma della precedente legge previdenziale. Analoga attenzione si è rivolta al tema del *welfare* sanitario, dedicando una misura specifica significativa

alle situazioni di svantaggio e di *handicap,* in nome di un principio di prossimità e di sussidiarietà che tiene insieme l'evoluzione del *welfare* pubblico con quello del *welfare* del privato sociale. Analogamente è stata confermata una misura di sostegno alla natalità, il cosiddetto *bonus* bebè, che nelle prossime legislature andrà accompagnato da una politica universale e organica sugli assegni ai figli e sul sostegno ai servizi alle persone. Infine, col fondo per il ristoro finanziario si è data una risposta concreta al dramma determinato dalla crisi delle banche. Voglio concludere con una rilevazione oggettiva. Noi ci sottraiamo alla forte *vis polemica* che abbiamo sentito in quest'Aula con due dati oggettivi. Alla senatrice Guerra, che ha citato una perdita di 2 milioni di unità di lavoro equivalente rispetto al 2008, ricordo che bisogna leggere i dati fino in fondo. Se noi rileviamo i dati dal 2013-2014, e cioè da quando è iniziata questa legislatura, i dati oggettivi rilevano una crescita di oltre 900.000 unità di lavoro equivalente in questo periodo.

o quasi unanime dei diversi Gruppi, che contrasta con lo spirito molto polemico che abbiamo sentito. Io vorrei riflettere per un attimo sui voti unanimi, perché ritengo abbiano un significato: esprimono la consapevolezza, anche da parte dell'opposizione, che, di fronte alla durezza delle sfide che ci attendono, esistono non risposte facili, ma assunzioni di responsabilità che per loro stessa natura sono sempre concretamente parziali. E sono però importanti perché - a nostro avviso - vanno nella giusta direzione, che è quella di creare sviluppo per poter creare lavoro lavoro e di poter disporre di risorse per favorire un *welfare* inclusivo e in grado di rispondere soprattutto alle gravi difficoltà

e con la legge di bilancio in esame rappresenti un ulteriore passo nella giusta direzione per le nostre famiglie, per il mondo del lavoro e le istituzioni democratiche, che offriamo alla valutazione dei cittadini. Intanto come Gruppo PD votiamo con convinzione il disegno di legge di bilancio e la fiducia al Governo.

i membri del Governo che hanno palesato delle esigenze e per coloro che hanno motivi di salute. Per il resto, mi dispiace ma non posso accoglierle.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.700 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 102-*bis* del disegno di legge n. 2960, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Onorevoli colleghi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.700 (testo corretto) gli articoli da 1 a 102-*bis* sono confluiti nel nuovo articolo 1 del disegno di legge. Avverto che i restanti articoli e i relativi emendamenti saranno comunque posti in votazione nella numerazione originaria, così come indicato nello stampato del disegno di legge. La Presidenza si intende fin d'ora autorizzata ad apportare le modifiche di coordinamento conseguenti all'approvazione dell'emendamento 1.700 Passiamo quindi all'esame dei restanti articoli del disegno di legge. Con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati, gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge. In questa fase della discussione, ai sensi dell'articolo 129, comma 5, del Regolamento, potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, e quindi il relatore e il rappresentante del Governo per esprimere il rispettivo parere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 104.Tab.2.5.5.

impegnati i Vigili del fuoco, in particolare quelli volontari, i quali sono particolarmente numerosi solo in una parte del nostro Paese, credo che sarebbe un riconoscimento veramente doveroso.

della conseguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile. La 5a Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea. In attesa della presentazione da parte del Governo della Nota di variazioni al bilancio, sospendo la seduta.

alle ore 21,18)*. Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018

ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, all'esame e alla deliberazione sulla Nota di variazioni, con la quale il Governo ha provveduto a introdurre nel testo del disegno di legge e nelle annesse tabelle le modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame degli articoli.

Signor Presidente, la presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 è stata predisposta al fine di recepire gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica al disegno di legge di bilancio. Tali effetti sono riflessi nella presente Nota di variazioni e sono neutrali rispetto agli obiettivi fissati nella manovra in termini di saldi di finanza pubblica. In relazione a quanto precede, la presente Nota aggiorna i valori contabili dell'articolo 16 (totale generale della spesa) del disegno di legge di bilancio e comporta modifiche: ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2018-2020 in termini di competenza e di cassa; allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle da n. 2 Si producono, in conseguenza, anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli. La presente Nota di variazioni, anche quest'anno, viene presentata secondo la nuova impostazione disposta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, che modifica la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009. Tale nuova impostazione discende dal fatto che, in base alle nuove disposizioni, i due disegni di legge che componevano la manovra triennale di finanza pubblica - disegno di legge di stabilità e disegno di legge di bilancio - sono ora integrati in un unico disegno di legge organizzato in due sezioni distinte. I prospetti per l'unità di voto e gli allegati tecnici per capitoli presentano ora l'intero bilancio dello Stato e non soltanto le unità e i capitoli che hanno subito variazioni per effetto degli emendamenti al disegno di legge. Le variazioni connesse agli emendamenti approvati sono esposte in apposite colonne distintamente per la Sezione I e la Sezione II. Passiamo dunque alla votazione della Nota di variazioni. Con l'approvazione della Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge, sia alle annesse tabelle.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 5 dicembre, alle ore 16,30, con all'ordine del giorno: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori». Sempre nella giornata di martedì, alle ore 13, è convocata la Conferenza dei Capigruppo